regolarmente convocato dal preside per qualche marachella che avevo combinato per essere processato, anche in quel caso, in direttissima. Le voglio dire che, comunque, avrei gradito almeno un avviso di garanzia,

stata una convocazione. È stata una richiesta, così come prevede il Regolamento, di poter fornire le proprie eventuali giustificazioni e osservazioni.

nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esamedell'articolo 36 concernente le disposizioni per la copertura finanziaria del disegno di legge. A seguito di alcuni rilievi emersi nel corso della discussione con riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 32, già esaminato recentemente, l'esame è stato sospeso per consentire alla Commissione bilancio di riunirsi per svolgere i necessari approfondimenti. In tale sede, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, è emersa l'esigenza di una proposta di coordinamento sulla quale è stata richiesta la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Chiedo quindi al presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, di riferire in merito alle determinazioni assunte dalla Commissione. un parere con il quale si richiede la riformulazione del comma 4 dell'articolo 32 nei termini che avevo anticipato questa mattina, che credo siano a verbale. Se i colleghi lo desiderano, posso rileggere il testo: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». Su questa proposta di riformulazione, abbiamo chiesto il parere della Ragioneria ed il Ragioniere generale dello Stato ha comunicato, con una nota firmata, che: «(...) è stato esaminato l'emendamento al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi, con il quale s'intende sostituire l'articolo 32, comma 4, relativo alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della delega prevista al citato articolo. Nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo occupazione, si concorda con le considerazioni svolte al riguardo dalla Commissione bilancio, ritenendo l'emendamento correttamente formulato». Per il resto, ovviamente la la competenza è di altri e non della Commissione bilancio. Signor Presidente, noi abbiamo stabilito, a mio parere, un principio assai pericoloso e cioè il fatto che questa Assemblea sia impermeabile a quello che accade all'esterno. Comprendo che questo principio non si possa mettere in dubbio, ma in ogni caso credo che sia doveroso da parte di tutti sapere che, nell'interruzione dei nostri lavori, c'è stata una dichiarazione del primo presidente della Corte Per favore, non interrompiamo chi sta parlando. Prego, senatore Quagliariello, Questi ha affermato di essere totalmente d'accordo con i rilievi critici che sono stati avanzati da altri ed in particolare dal presidente dell'Anac Cantone. Comprendo che questo dia fastidio e so anche che in altri tempi - lo dico agli amici ed ai compagni della sinistra - c'era chi diceva

tra le altre cose, di persone che hanno ruoli istituzionali, su un provvedimento di legge non ci sia mai stato. Mi rendo conto che questo non cambierà

tutto questo mi venga impedito e perché si debba ritenere non concedibile il termine per i subemendamenti a questa riformulazione della norma che stiamo discutendo.

e poi una proposta di coordinamento formale che riguarda l'articolo 32. Per quanto riguarda la proposta di coordinamento formale, essa fa evidentemente riferimento all'articolo 32, che è stato già votato dall'Assemblea. Quindi, il problema è comprendere se si tratti o meno di un vero e proprio coordinamento formale, oppure di una modifica del testo anomala rispetto alle regole che disciplinano il procedimento legislativo. Se non ho capito male, il presidente Tonini propone un coordinamento formale in virtù del quale la somma di 20 milioni di euro, originariamente stanziata nell'articolo 32, viene suddivisa in 7 milioni, 7 milioni e 6 milioni di euro nell'ambito del triennio. Personalmente, signor Presidente, credo che questo non possa essere considerato un coordinamento formale perché, ad esempio, ci potrebbe essere da parte di taluno l'idea di suddividere la somma di 20 milioni in termini diversi nel triennio, in ragione, ad esempio, delle previsioni di spesa

formale quanto proposto dal presidente Tonini. Conseguentemente, ove mai ciò dovesse accadere, vi sarebbe una violazione delle regole del procedimento legislativo. Pertanto, credo che la proposta di coordinamento formale non possa essere accolta perché fuoriesce dai limiti stabiliti dal Regolamento del Senato per il coordinamento formale e che, conseguentemente, la strada da percorrere debba essere necessariamente un'altra.

dal fatto che oggi ci vengono proposti un emendamento correttivo di quel coordinamento formale dell'articolo 36 e una nuova proposta di coordinamento formale

che ella stessa ha ritenuto di dover invitare i relatori a modificare in emendamento la proposta di coordinamento formale dell'articolo 36.

mentre l'articolo 32 è stato votato; essendo stato votato, non è possibile nessun'altra forma, se non quella del coordinamento. Naturalmente, quando affronteremo il problema della proposta di coordinamento, saranno affrontate anche queste questioni e l'Assemblea deciderà di conseguenza. L'emendamento 36.200 può essere votato, poi si voterà l'articolo; dopodiché, al momento delle proposte di coordinamento, si riproporranno queste questioni. Mi pare che la procedura sia chiara.

Il Presidente della Commissione bilancio, come suo solito, è stato preciso: questa è una riformulazione dell'articolo 32;

la si fa nella sede propria, ossia nell'altra Camera che prenderà prossimamente in carico il provvedimento. Così, penso di collaborare seriamente ad un'utile definizione di questi lavori.

Presidente. Lei sta seguendo l'obiettivo di trattare quella che è, come affermato dal Presidente della 5a Commissione, una riformulazione come una norma di coordinamento e all'osservazione avanzata dal presidente Azzollini ha risposto ha risposto che sia o no una norma di coordinamento, ne avremmo parlato dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale. Se al momento in cui dovessimo parlare della norma di coordinamento,

più pulita nel senso che se non facessimo così avremmo, dal punto di vista di una metà dell'Assemblea, una grave violazione del Regolamento dal punto di vista della maggioranza, la creazione di un precedente che, come qualcuno stamattina ha ricordato, potrebbe poi essere utilizzato al contrario negli anni che verranno. La cosa più opportuna, visto che al punto in cui siamo

ben si figura, in rappresentazione plastica, anche nella veste del suo Presidente, ed è per ammissione dello stesso Presidente che si è detto che forse c'è stata una dimenticanza. Come

rivotare una norma già votata. Questo ci farebbe incorrere in una grave violazione. Il modo più pulito di procedere, se siamo tutti d'accordo, è votare il provvedimento così com'è, tanto abbiamo già fatto delle variazioni e comunque il disegno

al suggerimento del Governo, come accortamente ricordato dal presidente Azzollini, possiamo benissimo trasformarlo in un ordine del giorno, questo caso all'unanimità, perché è una condizione *ex* articolo 81), dopo di che rivoteremo il provvedimento come ce lo rimanderà la Camera, nel modo in cui deve essere approvato per far sì che non incorra in problemi di incostituzionalità

come in questo caso. La riformulazione *ex* articolo 81 in questo caso non è stata fatta in Commissione bilancio, ma è stata proposta all'Assemblea e non è approvata con la giusta istruzione e la giusta presa

«La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo» quindi c'è un parere già espresso che integra il precedente parere «conferma il parere non ostativo con la seguente condizione,» quindi è un parere condizionato «ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata: specificata: "4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale

Presidente, recepiamo la proposta di coordinamento, facendo facendo presente, perché in questo senso va tecnicamente formulato, che il nostro emendamento si riferisce alle parti del comma 4 che vengono modificate, perché questa riformulazione non modifica integralmente il comma 4. Presidente, i relatori dicono che manterrebbero la loro proposta di coordinamento formale, facendo riferimento all'articolo 32 che abbiamo votato e che oggi diventa possibile modificare. A me sembra un po' fuori dal Regolamento, Presidente,

approvasse la richiesta, avanzata all'inizio di questa discussione dal presidente Romani, di ritornare in Commissione, tutto sarebbe possibile. Infatti, andiamo a ritoccare un testo votato e dovremmo votare se correggerlo secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

questo è pacifico. A questo punto, la tesi del presidente Azzollini, se non vogliamo tornare in Commissione, credo sia l'unica percorribile.

Questa è la proposta che viene fatta dai relatori, nel momento in cui hanno accolto il parere della 5a Commissione, come modificato e integrato rispetto al precedente.

ad una norma cosiddetta sovraordinata, come la legge n. 196 del 2009, in diretta dipendenza dalla norma costituzionale dell'articolo 81 e dalla n. Questo è il punto di fondo, per cui niente c'entra il coordinamento qui. Mi permetto di esprimerlo e ripropongo ciò che ho detto, proprio per consentire di andare avanti con regolarità.

lei ha messo in votazione qualcosa senza dichiarare cosa stesse mettendo ai voti.

non è che se mi prendo trenta secondi di tempo, con tutti i discorsi inutili che facciamo, lei mi deve riprendere sempre dicendo che stiamo perdendo tempo:

(al di là di tutti i problemi e le riserve che abbiamo sulla possibilità che questo venga fatto attraverso un coordinamento, dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale), se ha già sottoposto al voto l'emendamento 36.200 contraddice questo assunto. Infatti, già mette al voto una parte di coordinamento, che è quella che potrebbe essere intesa davvero come più di coordinamento dell'altra; dopo di la parte che non è di coordinamento (e che sarebbe meglio fosse assorbita in questa proposta di coordinamento) lei la propone come coordinamento. Che motivo c'è di mettere al voto questo emendamento

questo come un parere e così l'ha trattato, chiedendo ai relatori il parere sulla proposta, ma non c'è un parere dei relatori sulla proposta. Quando viene fuori dalla Commissione bilancio un parere contrario *ex* articolo 81 questo deve essere messo all'interno del testo votato, altrimenti, se non si mette all'interno del testo votato, il testo che si vota è invotabile perché contrario all'articolo 81. Quindi, non c'è un parere ed è una correzione sostanziale dell'impianto dell'articolo 32:

chiedo scusa - di pensare che questo le fosse stato chiaro, visto il mio precedente intervento e che glielo avessero chiarito gli uffici. Per questo le ho domandato se stessimo votando

di prendere il nostro come un consiglio, lo si prende soltanto con spirito e vena polemica e come un tentativo di fare ostruzionismo. Di questo, se mi permette, un po' mi dispiaccio ed ecco perché poi alzo i

Ho già richiamato stamattina il parere della Commissione bilancio che imponeva la cancellazione del quarto comma (allora sesto)

*ex* articolo 81 della Commissione bilancio, quindi, l'articolo 113*-bis*, comma 4, o si mette qua o non c'è coordinamento e, sotto il profilo della correttezza del procedimento legislativo, quella è una violazione.

L'articolo 32 - lo dico per chi non lo ricordasse - è interamente di coordinamento: è stato dettato dalla Commissione bilancio e trasformato in emendamento dai relatori.

votato dall'Assemblea e che era della Commissione bilancio. Quando l'avremo votato, lei mi dirà che dovremmo porci il problema se l'articolo 32 è corretto o meno ed è una questione di lana caprina, peggio di quella dell'articolo 27, perché lì abbiamo la certezza matematica, che è tranciante, dell'articolo 81. Qui, invece, abbiamo un testo votato, su suggerimento della Commissione bilancio, e tutto

Per quanto riguarda l'articolo 32, credo che se votiamo questo emendamento non abbiamo risolto il problema, perché non potremo votare una correzione dopo il coordinamento.

Cerco di spiegarmi: *errare humanum est, perseverare autem diabolicum*, e noi l'articolo 32, non solo lo abbiamo votato, abbiamo rivotato in questo momento. Allora, qualcuno mi vuole spiegare, dopo aver votato due volte il medesimo articolo, come diavolo si fa a inserire una norma di coordinamento? Perché, secondo me, a questo punto la legge muore? Perché, a questo punto, il coordinamento proposto dalla Commissione bilancio è una condizione obbligatoria affinché la legge sia Ma, nel momento in cui dovessimo votare quella norma di coordinamento, noi andremmo

Signor Presidente, colleghi, prendo la parola a nome della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto per esprimere il nostro voto favorevole a questa importante riforma del codice antimafia. Voto favorevole che esprimiamo, non solo e non soltanto perché si è preso un formale impegno, da parte del Governo e della maggioranza, con l'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma del a procedere a mettere mano all'articolo 67, comma 6, del testo unico antimafia per riportare la cosiddetta legge Lazzati alla sua originaria formulazione, così da impedire finalmente ai sorvegliati speciali per mafia

Come Italia dei Valori esprimiamo voto favorevole, non solo per questo, ma soprattutto perché questa riforma porterà a una migliore efficienza dell'operato attraverso l'Agenzia dei beni confiscati, grazie sia alla sua riorganizzazione, che all'aumento della dotazione del personale, soprattutto perché si procederà alla valorizzazione effettiva dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, affinché il contrasto sul piano patrimoniale sia reale.

tale e quale, in questa legislatura e che è entrata a far parte di questo disegno di legge. Nella legge di iniziativa popolare si richiedeva che i patrimoni sottratti alle mafie ritornassero utili al bene comune, così da poter finalmente utilizzare gli oltre venti miliardi finalizzandoli allo sviluppo e al lavoro, infliggendo un grande dolore alle mafie che soffrono, come gergalmente si usa dire, per i "piccioli" che vengono loro confiscati. Questa riforma rappresenta lo strumento fondamentale per il contrasto effettivo alle mafie in quanto accelera il procedimento giudiziario che dal sequestro porta alla confisca definitiva dei beni mafiosi, consentendo alla comunità di poterne usufruire in tempi più celeri. Ancora, votiamo favorevolmente pur consapevoli delle criticità presenti sul lato dell'estensione delle misure di prevenzione anche ai reati non direttamente collegati al 416-*bis*, cioè mafiosi, a cominciare dai delitti commessi dai corruttori, passando per i reati collegati al terrorismo

prefetto Gabrielli ha riportato che ultimamente è diminuita la percentuale di donne uccise. È pur vero che il numero rimane molto alto, per cui anche questo correttivo all'interno del codice antimafia potrà aiutare a prevenire questo odioso reato.

per la verità questa mattina abbiamo sentito in Commissione accusare i colleghi e il Senato in generale

della normativa antimafia per quanto riguarda i sequestri e le confische anche a tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Vorrei allora mostrare ai colleghi, a chi ci ascolta e a chi ci

Giovanardi dichiara: «Ai miei occhi» l'articolo 1 «è demenziale. Sarà sufficiente essere indagati» - adesso sappiamo che è sufficiente un indizio «per corruzione e un giudice potrebbe sequestrare un intero patrimonio» e naturalmente, avendo esteso a più di trent'anni la prescrizione, dopo la confisca si dovranno aspettare anche trent'anni per sapere se si è colpevoli o innocenti. Pertanto, non solo ci eravamo accorti di quello che stava accadendo, ma l'abbiamo denunciato fortemente, purtroppo purtroppo senza ricevere una grande attenzione mediatica sulla denuncia e sulla gravità di quello che sta accadendo, nel momento in cui si annacqua la normativa antimafia allargandola a tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

scolpito in difesa della dignità di ogni singola persona e di un diritto penale che colpiva persone che avessero compiuto un determinato reato. modo al fascismo: Dino Grandi disse, in occasione della riforma del codice penale, che non devono esistere «confini o diaframmi tra politica e diritto, ma siamo convinti che fra essi vi sia invece un nesso assoluto in quanto rappresentano fasi indissociabili nel divenire di un popolo». Quindi, dal punto di vista del fascismo, c'è la subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività nazionale. E non a caso fu proprio il fascismo a rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione, che prescindono dal sistema retributivo delle pene fondate sul fatto. Ebbene, qui stiamo parlando di confisca di beni senza che ci sia non una sentenza passata in giudicato, ma neanche un rinvio giudizio. giudizio. Il nazismo, nel suo codice penale, prevedeva la stessa cosa e cioè che: il giudice, violando i principi di legalità e di retroattività - come facciamo noi con questa legge e il principio di applicazione analogica, potesse punire una condotta sulla semplice base della sua contrarietà al sano sentimento popolare: chi contrasti il sano sentimento popolare può essere condannato. Nel codice penale sovietico poi, c'era il famigerato articolo 58, con 14 commi talmente omnicomprensivi - come spiegò Solženicyn in «Arcipelago gulag» - che qualunque attività svolta da qualsiasi persona poteva essere definita controrivoluzionaria se diretta a sovvertire o indebolire il Consiglio dei lavoratori, la sua sicurezza o i guadagni della rivoluzione proletaria. Anche qui c'era la confisca dei beni beni (e la pena di morte in alcuni casi) per la cosciente non esecuzione o deliberata imprudenza nel compiere i propri doveri con lo scopo di sabotare le attività statali. Come vedete, niente di nuovo sotto al sole. Stiamo tornando ad una regressione del diritto penale tipica dei regimi totalitari, con le stesse motivazioni che abbiamo sentito sostenere nei regimi totalitari. Questa volta è la corruzione dilagante. Quale? Quella dei sondaggi di opinione? Più volte ho detto in quest'Aula che ci sono 300 processi processi all'anno per corruzione nel nostro Paese che non finiscono in prescrizione ma, secondo i sondaggi di opinione, l'Italia è all'ottantesimo posto tra i Paesi più corrotti del mondo. Sarebbero milioni, sempre secondo i sondaggi, le persone italiane che si vedono chiedere tangenti e nell'ultimo sondaggio, siamo arrivati a 160 miliardi di tangenti ogni anno. Prima erano 60 miliardi, adesso siamo a 160 miliardi, cioè, italiana, siamo a due miliardi di tangenti, quindi, saremmo un popolo fatto soltanto di corrotti e corruttori, compresi coloro che dovrebbero combattere la corruzione. Questa è la diagnosi che viene fatta per poi portare avanti questa drastica terapia. Mi domando, allora, e continuo a dirlo: non è che forse qualcuno è interessato a buttare a mare tutta la strumentazione efficace contro la mafia, che sono leggi eccezionali che però hanno superato il vaglio della Corte costituzionale e anche dei tribunali europei proprio per la specificità e la pericolosità della 'ndrangheta, della mafia e della camorra?

Nessuno si pone questo problema? Usciamo dalla Costituzione, imitiamo i regimi totalitari, spariamo con il cannone contro realtà assolutamente variegate e poi bisognerà andare a spiegare ai sindaci, agli assessori

andiamo contro il diritto europeo, imitiamo i sistemi totalitari, provochiamo smarrimento in chiunque abbia un po' di buon senso nell'andare a fare l'amministrazione pubblico perché stiamo stabilendo

Poi vedo che, malgrado tutto questo, non si riesce a ragionare in termini di quello che andava bene a tutti. Il 90 per cento dei componenti di questo Parlamento, compreso il sottoscritto da quando è qui, ha sempre votato tutte le norme di rigore contro la mafia: le leggi eccezionali, il carcere duro, tutto quello che volete. Sull'affinamento della gestione dei beni confiscati ai mafiosi, onde evitare che finiscano in circuiti circuiti opachi o di cattiva gestione, c'è stata unanimità in Commissione, quindi questo è un provvedimento che poteva uscire da quest'Aula come un segnale forte di tutto il Parlamento quattro la criminalità organizzata. Mi spiegate perché qualcuno, invece, ha avuto l'idea, nell'articolo 1, di estendere le misure anche ai reati contro la pubblica amministrazione? Chi ha avuto quest'idea? A chi serve? Ai magistrati? Dicono di no. A chi combatte la corruzione? Dicono di no. Ai Presidenti emeriti della Corte costituzionale? Dicono di no. Alle camere penali e a tutti gli avvocati? Dicono di no. A chi serve

usciamo invece divisi, con una norma sbagliata, di cui naturalmente i proponenti risponderanno davanti al Paese, anche in termini di violazione gravissima della nostra civiltà giuridica.

una volontà unitaria di adottare norme serie per combattere un fenomeno così difficile e pericoloso quale quello mafioso.

invece portato avanti il lavoro quasi a voler mettere delle toppe continue rispetto a rilievi e a perplessità che sono state considerati anche in Commissione e che fortunatamente alcuni membri della Commissione hanno sollevato, altrimenti ci sarebbero stati anche degli errori macroscopici. Purtroppo, però, per affrontare la mafia occorrono decisione

che fu combattuto con armi pesanti, che sono leggi e che devono essere delle leggi particolari.

Questa è una delle grandi problematicità che sono emerse, che è apparsa chiara a tutti i colleghi: è vero che il Parlamento deve essere principe nell'elaborazione e nell'emanazione di una legge e che deve essere il più possibile non influenzabile, ma non possiamo non tenere in considerazione i rilievi che sono stati sollevati.

volte la lotta alla mafia sembra quasi un argomento retorico, mentre si deve pensare alla gravità effettiva del fenomeno e di come esso si è evoluto nel tempo. Ormai non si pensa più all'immagine del mafioso con la coppola e la lupara,

Mi riferisco peraltro ai colleghi che hanno lasciato l'Aula, mostrando poco interesse alla discussione di un tema così delicato. L'impianto delle misure di prevenzione,

hanno ben capito questa cosa. Molti Paesi ci hanno anche un po' scopiazzati, invidiandoci il coraggio il coraggio di aver realizzato un sistema di prevenzione che vada a colpire la criminalità organizzata e le mafie prima ancora che si accerti la responsabilità. Se il sistema penale italiano per essere funzionante deve necessariamente passare non già attraverso un processo, ma attraverso tutte quelle misure cautelari (vedi anche queste), da operatore del diritto mi sento alquanto scoraggiato.

ha acquisito una certa cultura rispetto a un provvedimento che va a intaccare quel sistema e l'impianto di quelle misure di prevenzione). prevenzione). Probabilmente, il danno maggiore che arrecate con questo provvedimento

nell'affermare la bontà delle misure di prevenzione, quando venivano rivolte alla criminalità organizzata. Questo è quanto, sotto il profilo squisitamente tecnico. C'è ancora da rilevare a questi miei colleghi, uditori assenti,

Abbiamo esteso le misure di prevenzione ai reati contro la pubblica amministrazione. In un primo momento, in discussione generale feci notare che avevano inserito anche il peculato d'uso, cioè un amministratore che utilizza l'auto per fini personali andava incontro alle misure di prevenzione, quelle personali ed eventualmente quelle patrimoniali. Questo aspetto è stato corretto stato corretto ed eliminato. È stato creato un collegamento con l'articolo 416 del codice penale ed è stato lasciato fuori il reato di truffa aggravata,

la truffa aggravata è delitto che si consuma generalmente in concorso con altre persone, tant'è che mi presi la briga di andare a guardare il repertorio della giurisprudenza penale e portai in le sentenze che vedevano condannato un solo individuo per il delitto di truffa aggravata. Avevo chiesto - gridando - di permetterci di votare. Noi non possiamo non possiamo non votare un provvedimento di contrasto alla criminalità organizzata e non possiamo non farlo per la nostra storia. Infatti la storia di chi siede da questa parte dell'Aula è segnata da provvedimenti che hanno contrastato fortemente la criminalità organizzata. Il carcere duro, ma anche le attuali misure di prevenzione, sono provvedimenti che sono stati emanati delle forze di centrodestra di questo Paese, ed oggi si impedisce a queste stesse

Non è un provvedimento che, al di là del titolo, sortirà effetti di contrasto alla criminalità organizzata. Non è un Non è un provvedimento che contrasta, anzi, non so prevedere il futuro ma sono convinto che questa estensione comporterà necessariamente l'incostituzionalità di tutto il sistema e ci ritroveremo a non poter utilizzare neanche per i mafiosi l'efficace strumento delle misure di prevenzione. Ho detto che

che farcene, non ricorriamo a questo genere di professionisti, miriamo alla sostanza delle cose e in questo provvedimento la sostanza non c'è.

ci apprestiamo a dare il via libera definitivo per questo Senato alle nuove norme in materia di misure di prevenzione e, in particolare, in materia di codice antimafia e antiterrorismo. Nonostante la vulgata e la necessaria semplificazione giornalistica, non si tratta di norme da far valere soltanto nel contrasto alla mafia, ma di norme che incideranno in maniera profonda e sostanziale nel contrasto a varie forme di criminalità e che si pongono l'obiettivo di aggredire il fenomeno criminale subito, al suo primo apparire: non *ex post* (cioè a delitto compiuto), ma *hic et immediate*, per quanto possibile, con la finalità e nel tentativo di precedere (come criterio di prevenzione generale) e di prevenire, nello specifico, la consumazione piena dei più gravi reati e comunque di impedirne la protrazione ed il godimento. Esiste nella nostra società e nella classe politica, come abbiamo visto anche durante i nostri lavori d'Aula, una sorta di schizofrenia e al contempo di comportamento farisaico. Non si può infatti, da un lato, chiedere sicurezza sociale e individuale, pretendere giustamente il rispetto dei principi processuali penali costituzionali e, dall'altro lato, subito dopo, di fronte a fenomeni criminali caratterizzati soprattutto dalla pervicacia e dalla recrudescenza, tanto da destare serio e fondato allarme sociale, cercare in ogni modo di impedire che questi fenomeni vengano adeguatamente aggrediti, prima che siano portati alle estreme conseguenze, con le forme e gli strumenti delle misure di prevenzione o di sorveglianza, già previste dal nostro ordinamento, per ogni tipologia di delitti, anche meno gravi di corruzione e concussione, a determinate condizioni. Va ricordato infatti che il sistema delle nostre misure di prevenzione, nel suo insieme, è un sistema che è già in vigore, rodato e che funziona da anni. È un sistema che ha ripetutamente passato il vaglio severo della Corte di cassazione, della Consulta italiana e delle Corti di giustizia europee. È indubitabile però la necessità di un aggiornamento e di una rimodulazione di questo sistema, alla luce sia dell'esperienza maturata, con particolare riferimento alla gestione dei beni e delle aziende sequestrati, sia della maggiore sensibilità nei confronti di nuove evenienze ed emergenze criminali. Se è meno complicato trovare un accordo politico ampio nella lotta al terrorismo, particolarmente internazionale, già più complicato appare giungere ad un consenso politico in ordine a sistemi preventivi e più efficaci nei confronti del crimine mafioso. E se tanti blaterano, a parole, contro i gravi scandali sul fronte della corruzione, molti di meno sono coloro che cercano, realmente e concretamente, degli strumenti per contrastare alla radice, oltre che culturalmente e amministrativamente, ogni apparizione, già *in nuce*, del corrotto, del corruttore, del concussore. E pur facendo sempre salvi le finalità, le regole e i tempi del processo penale, che è però un processo per sua stessa natura repressivo, ma postumo, "a babbo morto" si direbbe. E ancor più delicata è la situazione delle vittime di *stalking*. Quante volte abbiamo sentito criticare, anche aspramente, la polizia e la magistratura per non essere intervenute tempestivamente a tutelare una donna, in inesorabile successione temporale, aggredita, violentata e magari trucidata? E quante volte si è risposto che le norme sostanziali e procedurali sugli atti persecutori non lo consentivano? O magari sono sbagliate, come l'ultima approvata votando la recente riforma del codice penale? Ora, il Parlamento non si può girare dall'altra parte. È compito del Parlamento provvedere e oggi è compito di questo Senato, approvando questo disegno di legge, decidere di impedire e ostacolare da subito la consumazione anche di questo crimine particolarmente odioso. Nessuno si vuol nascondere dietro a un dito e nessuno vuol negare che, per alcune norme, si viaggia sul filo della legittimità costituzionale, ma all'interno di questa legittimità. Ma solo su una norma - lo sottolineo: soltanto su una norma - solamente ora si discute animatamente; si è scatenato addirittura un putiferio sulla norma che estende a corrotti e concussori, in forma peraltro temperata, le misure di prevenzione. Sarebbe da chiedersi il perché. La norma ci era arrivata dalla Camera dei deputati in una formulazione molto più ampia, pressoché totale; in Senato è stata corretta e qualche solone critico non se ne è nemmeno accorto, accorto, ed è stata resa più stringente e collegata al reato associativo, rispondendo proprio alle ricordate necessità fattuali, logiche e giuridiche,

se il rispetto dei parametri costituzionali sarà soddisfatto anche dalla nuova previsione relativa ai delinquenti corrotti associati, da sottoporre a misure di prevenzione, o se il legislatore dovrebbe fermarsi a prevedere queste misure solamente per mafiosi e terroristi. In ogni caso si tranquillizzino i novelli oracoli dell'antimafia e dell'anticorruzione interni ed esterni a quest'Aula, perché le due fattispecie di previsione sono autonome e da nessuna parte sta scritto della loro inscindibilità. Non vige in questo caso il principio del *simul stabunt, simul cadent*. Con il provvedimento oggi al nostro esame, invece, che è molto più ampio e con molte altre norme certamente positive, in primo luogo si vorrebbe intervenire per regolare, registrare e adeguare alla fenomenologia criminale odierna alcuni istituti giuridici già esistenti nel nostro ordinamento, in materia di lotta alla grande criminalità e al terrorismo, come ad esempio in tema di sequestro e confisca dei beni e in particolare dei patrimoni, non solo per reati di mafia, ma anche per il caporalato, per i cosiddetti ecoreati e per il riciclaggio. Più nello specifico, si vuole intervenire sulla *vexata quaestio* dell'amministrazione, della gestione e della destinazione di tali beni sequestrati e confiscati, oltre che sul controllo giudiziario delle aziende e sugli strumenti finanziari e di premialità fiscale e contributiva, necessari per assicurare l'efficacia e la sostenibilità delle aziende sequestrate e confiscate.

sulla scia di quanto già previsto nel disegno di legge per gli amministratori giudiziari dei beni sequestrati. In secondo luogo, si interviene sia per confermare la platea dei destinatari delle misure di prevenzione personali e reali, anche relativamente ai fatti di terrorismo e di eversione, sia per prevedere un allargamento della platea di questi destinatari a persone implicate formalmente in fenomeni delittuosi, che la nuova e più recente sensibilità sociale e politica ritiene di dover sottoporre, non solo a processo penale, ma pure ad adeguati e moderni sistemi di prevenzione. Mi riferisco, in maniera chiara e come già accennato, all'elenco di reati e di soggetti destinatari, di cui agli articoli 4 e 16 del testo così come da noi modificato, pur tra tante polemiche e contestazioni da parte della destra politica. Ciò significa che, d'ora in poi, soggetti destinatari delle misure in questione saranno non solo i mafiosi o i terroristi,

che sottolineano la necessità di tutela prima che il delitto possa essere portato alle più deleterie e nefaste conseguenze). Soggetti destinatari delle misure sono, ancora, i corrotti, i corruttori e i concussori nell'ambito di una associazione a delinquere, così come coloro che mettono in pericolo l'incolumità pubblica, anche in occasione o a causa di manifestazioni sportive,

Anche in tema di lotta alla corruzione, una delle più gravi e annose emergenze sociali, amministrative e politiche della nostra società, come continuano a ripeterci pure tutti gli osservatori indipendenti sia nazionali che internazionali, oltre che tutti gli organismi italiani di controllo istituzionale in materia (tanto che si ritiene di dover parlare di una vera e propria piaga nazionale), questo disegno di legge interviene in maniera chiara e netta, nel rispetto della legalità costituzionale e dando in modo deciso l'idea di un legislatore che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della corruttela, sì dal punto di vista della repressione, ma soprattutto dal punto di vista della prevenzione, sia generale che speciale. E confermando l'idea che la corruzione va combattuta sotto ogni punto vista, facendo in modo che essere corrotti o corrompere non paghi nemmeno più: far venir meno, infatti, per la corruzione il substrato e il conseguimento di interessi economici, finanziari e di ogni sorta di profitto, come per i delitti di mafia o di truffa aggravata, farebbe venir meno il senso stesso del delinquere, finalizzato alla ricerca e acquisizione del profitto illecito.

da interventi nella logica dell'azione dopo che i buoi sono scappati dalla stalla lasciata aperta, a interventi lungimiranti e mirati alla tutela preventiva dei nostri beni e dei nostri valori, nel rispetto sempre della Costituzione. Quei valori che vuole salvaguardare questo disegno di legge: l'integrità fisica e morale delle persone, la tutela delle vittime dei crimini di terrorismo, di mafia, di *stalking*, di concussione, il rispetto della legalità, la difesa del nostro ordinamento costituzionale. Per tutti questi motivi e per dare un segnale forte e chiaro di lotta a tutte le mafie e alla corruzione, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e

Vorrei provare a dare una ricostruzione temporale del provvedimento in esame e forse riuscirò a dare anche qualche risposta al collega Giovanardi del perché dello stesso. Questo provvedimento Questo provvedimento viene licenziato nel 2015 dalla Camera dei deputati e poi non ci vuole molto: ho imparato in questi quattro anni che il provvedimento può rimanere tranquillamente nei cassetti e infatti ci rimane per due anni e a un certo momento diventa molto urgente, e la cronaca di questi giorni di come si è sviluppato il dibattito in Aula si incaricherà di dimostrare quanto arruffato sia il provvedimento stesso. Perché allora a

tendono ad arrivare a delle conclusioni. Mi piace riuscire a parlarne oggi perché la "levata" di quella interrogazione del senatore Zanda contro la procura di Napoli e contro

questo pare se ne sia reso conto anche un certo Vittorio Tutino, che non è uno qualsiasi: è un *boss* palermitano di cosa nostra che è stato assolto dall'accusa di aver preso parte alla strage di Capaci ed è imputato per la strage di via D'Amelio. Ragionando sulla situazione attuale di contrasto alla mafia Vittorio Tutino afferma: «Non sono più i tempi in cui Berta filava». Signor Presidente, lungi da me il credere che Vittorio Tutino conosca la storia di Bertrada di Laon,

e che il tanto conosciuto e vituperato 41-*bis* è annacquato da discutibilissimi provvedimenti amministrativi, che denunciano un sistema carcerario ormai fuori controllo e non più sotto il governo dello Stato.

ne approfitto anche per perpetuare gli insegnamenti di un fratello magistrato la cui memoria viene oggigiorno infangata e vilipesa da una conventicola di magistrati i quali difettano buone nozioni di diritto e buone pratiche di polizia giudiziaria, ma non certamente di spiccate doti di fantasia e di palcoscenico mediatico. Cos'è questo Nasce per impedire ai detenuti mafiosi di comunicare all'esterno ordini e messaggi. Il regime carcerario previsto da questo articolo, nonostante, come detto, l'irrigidimento, va via via perdendo la sua efficacia a causa di pratiche consolidate che ne svuotano l'originaria funzione. Come è stato rilevato dalla Commissione antimafia, si sta assistendo a una pericolosa prassi che viola il divieto sancito dall'articolo 41*-bis* di contatti dei detenuti con l'esterno. Penso, ad esempio, ai permessi eccezionali accordati ai *boss* per le visite ai propri familiari.

che vengano garantiti determinati servizi all'interno delle carceri e che, ai soggetti ai quali si applica il 41-*bis*, sia data la possibilità di utilizzare Skype. E sia, andiamo avanti così! ci sono anche casi eccezionali cui vengono accordati permessi. Penso, per esempio, a Salvatore Pesce, arrestato nel 2011 e sottoposto a 41-*bis* proprio a causa della sua forte *leadership* criminale nel territorio calabrese. Pesce è stato autorizzato a tornare proprio in quel territorio con tanto di scorta della polizia penitenziaria. Il risultato è stata un'interminabile processione di persone che si sono recate in pellegrinaggio davanti alla casa del *boss*. Non è questo l'unico caso. Questi casi avvalorano quanto affermato dal *boss* Tutino. Nel 1992, anno di produzione della norma, sino al 2009 nessun permesso di tale tipo era stato mai concesso. assistiamo a un preoccupante incremento del fenomeno. Dall'inizio di questo anno i magistrati di sorveglianza hanno disposto, sulla base di emergenze rappresentate dai detenuti, 17 permessi, che, tra l'altro, costano ai cittadini circa 20.000 euro ciascuno. Lo scorso anno sono stati 20 i detenuti riportati a casa e la cronaca di oggi si incarica anche di dirci che, usufruendo di questi permessi, autorevoli esponenti del mondo della criminalità possono darsi alla latitanza. Non solo, in nome di un garantismo di maniera, avallato dalle miopi scelte di politica giudiziaria della maggioranza e del Governo, siamo costretti a vedere assestati ulteriori colpi a quel regime carcerario duro che voleva spezzare le relazioni dei mafiosi con famiglie e territorio. relazioni la mafia ieri ha fatto esplodere mille chili di tritolo, mentre oggi si va rinsaldando senza alcun rumore grazie alla prassi della trasformazione del regime del 41-*bis* in alta sorveglianza per i detenuti mafiosi. Direte: ma il codice antimafia? Credo che le vicende del 41-*bis* siano emblematiche. Ne parlo perché ho l'impressione che questo provvedimento non tenga adeguatamente conto di elementi essenziali di un'efficace normativa antimafia, segnalati del resto da primari soggetti istituzionali quali la Commissione antimafia e la procura nazionale antimafia, Stando così le cose, le istituzioni stanno allentando la presa oppure si sta sviluppando un'interpretazione della norma che comunque ottiene il risultato di un minor rigore che, a sua volta, ingenera l'idea di una logica di favore? Ovviamente tutti siamo d'accordo sulla necessità di perseguire una lotta dura alla mafia. Dunque, sarebbe stato opportuno eliminare ogni margine di discrezionalità, utilizzando i dati acquisiti e le osservazioni espresse proprio dalla Commissione antimafia, così da riscrivere una norma che meglio avrebbe garantito l'originario spirito dell'articolo Un altro esempio che a me pare significativo dei possibili interventi migliorativi di un testo che risulta asfittico concerne la salvaguardia del valore dei beni sequestrati ai confiscati. Sono anni che si parla di questa problematica, ma ritengo che i contenuti del testo approvato in Commissione si muovano ancora in una ottica troppo burocratica e procedurale, piuttosto che affrontarne gli aspetti concreti. È dato comune, infatti, che molti (secondo me troppi) dei beni oggetto di misure patrimoniali finiscono per perdere il loro valore. Ciò riguarda in modo particolare le aziende. Si tratta di beni che richiedono necessariamente modalità di gestione che ne consentano, sin dalla fase del sequestro, la salvaguardia del valore ovvero della loro capacità produttiva. obiettivo che consentirebbe di perseguire sia l'interesse del titolare dell'azienda in ipotesi di esito favorevole del procedimento penale a suo carico, sia della collettività in caso, invece, di esito negativo del procedimento stesso, collettività che potrebbe avvantaggiarsi da un bene sequestrato gestito con criteri di economicità e di mercato, contrariamente a quanto di fatto continua ad accertare, nonostante una normativa che vorrebbe perseguire proprio quell'obiettivo. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, importanza, ancora una volta, nonostante le buone intenzioni, mi sembra che il provvedimento evidenzi una scarsa attenzione agli aspetti garantistici del procedimento di prevenzione. Un procedimento, disegnato dal testo che stiamo licenziando, che temo non tenga in adeguata considerazione tale fondamentale aspetto, quello delle necessarie garanzie difensive, che dovrebbe essere il *fil rouge* che lega tutta la normativa procedimentale in quanto queste garanzie sono connaturate con le fondamenta dello Stato di diritto (ci siamo spellati le mani l'altro giorno nel ricordare Rodotà e questo argomento).

le misure di prevenzione nei confronti degli *stalker*, che sono state ben ricordate sia dalla senatrice Ricchiuti che dal senatore Casson, gli elementi che ho ricordato continuano, secondo me, a dimostrare un fatto fondamentale: questo provvedimento è fatto solo per poter essere utilizzato in campagna elettorale e noi non possiamo continuare a legiferare nel tentativo di dare delle risposte all'opinione pubblica che vanno nell'interesse del Partito Democratico. Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo GAL voterà contro questo provvedimento. Signor Presidente, cercherò di essere il più sintetico possibile. L'obiettivo principale di questo disegno di legge è ben distante da tutte le questioni poste in Aula, per come ordinariamente capita allorquando il dibattito diverge su questioni che non colgono l'essenza, la cosa più importante. D'altronde, una riforma a distanza di pochi anni dall'introduzione del codice antimafia non si giustificava se non si fosse colto un aspetto davvero fondamentale. L'aspetto fondamentale da correggere è costituito dalla gestione dei beni, soprattutto allorquando si tratti di aziende. È bene dire che l'obiettivo principale di questo disegno di legge è consentire che le aziende costituiscano una opportunità economica per la collettività, e, allorquando al sequestro non consegua la confisca, siano restituite a coloro i quali ne hanno diritto nelle medesime condizioni nelle quali esse erano state sequestrate. Il disegno di legge, dunque, coglie un obiettivo essenziale: il contrasto alla criminalità organizzata si vince anche se lo Stato si presenta come soggetto in grado di distribuire benessere, di garantire il mantenimento dell'occupazione, allorquando l'occupazione c'è e, quindi, se coglie l'obiettivo di consentire che queste aziende partecipino alla composizione del PIL nazionale. Noi abbiamo fatto di tutto in questa direzione; abbiamo anche scritto un secondo codice antimafia (è bene dirlo, in un contesto nel quale non è nemmeno riconosciuta l'importanza delle cose fatte). Noi pensiamo di avere contribuito in questa direzione; forse avremmo voluto fare di più, e chi conosce le tante traversie che la discussione del disegno di legge ha dovuto attraversare, comprende il senso delle frasi che sto pronunciando. Quindi questo era il vero obiettivo della riforma. Ripeto, cogliere questo obiettivo significa presentare lo Stato non come un liquidatore che interviene per dismettere attività produttive, ma come un soggetto che, interrotto il rapporto di dipendenza con la criminalità organizzata, ciononostante utilizza in senso economico e nell'interesse collettivo queste aziende. Questo è il primo punto sul quale abbiamo speso il nostro impegno. che questo disegno di legge è stato tenuto nel cassetto per due anni, non conosce il volume di lavoro che è stato svolto e forse non gli interessa conoscerlo, in un'epoca della *post*-verità, nella quale la verità senza ogni altra qualificazione non interessa a nessuno, mentre a tutti interessano le congetture, le illazioni, se non addirittura le chiacchiere. Questo è il primo punto. C'è un secondo punto del quale voglio parlare ed è un tema storico: quello del garantismo. Il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione è un processo non garantista, bensì sintetico. Perché è sintetico e non garantista? Perché le misure devono avere una funzione soltanto preventiva. È chiaro - e qui mi indirizzo a tutti i senatori presenti - che, se noi superiamo questo parametro di prevenzione e quindi debordiamo verso misure punitive, il codice si espone a quei rischi di costituzionalità con i quali devo dire tardivamente - e sottolineo tre volte l'avverbio si è discusso in questi giorni, dopo che la Commissione di questi problemi si era fatta carico. Se ne era fatta carico concretamente, non soltanto perché noi sappiamo dell'uomo era intervenuta con la nota sentenza De Tommaso (della quale ovviamente nessuno ha parlato), con la quale alcuni aspetti delle misure di prevenzione venivano in un certo senso accusate di violazione delle regole della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. per rispondere a questo dubbio di costituzionalità del processo per l'applicazione delle misure di prevenzione, avevamo proposto una serie di innovazioni, che non avrebbero ovviamente colmato la differenza che separa il processo ordinario da quello di prevenzione, ma avrebbero reso il processo di prevenzione più garantito, più protetto rispetto a quei rischi di costituzionalità dei quali - ripeto l'avverbio - tardivamente, molto tardivamente si è parlato. Tra le tante cose che siamo riusciti ad introdurre - io avrei voluto molto di più in questa direzione - vi è il diritto alla prova, che costituisce un'innovazione del tutto rivoluzionaria - uso un termine pregnante, consapevole del significato che gli va attribuito

questo emendamento che noi abbiamo voluto e che abbiamo presentato, fortunatamente - e anche qui utilizzo un avverbio pregnante - è passato, ma di ciò nessuno si è accorto. Anche i tanti interventori postumi distratti non si sono accorti che il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione, seguendo le indicazioni di una nota sentenza a sezioni unite (la è cresciuto quanto a livello di garanzie e quindi è maggiormente protetto dai rischi di incostituzionalità. Concludo - perché è stato l'unico emendamento che ho presentato a mia firma con questa introduzione: io credo che salverà qualche vita; e se anche ne dovesse salvare una sola, il Senato sarà orgoglioso di essere stato protagonista di un tentativo reale di proteggere tante vite di giovani donne sventurate che vengono uccise, con una reiterazione di condotte che costituisce un problema davvero allarmante sul versante anche della coesione della nostra società. Ho inteso proporre - poi, ovviamente, la Commissione e l'Assemblea hanno conseguentemente votato - una norma che non contraddice la struttura sistematica delle misure di prevenzione, perché lo *stalking* è un delitto che implica condotte reiterate e, quindi, siamo nel sistema delle misure di prevenzione; ma poi, sulla base anche della consapevolezza - si è ritenuto di introdurre che la norma di cui all'articolo 612-*bis è* indimostrabile in giudizio. Questo è un discorso costituzionale, perché la Corte costituzionale ne ha parlato a proposito del delitto di plagio: troppe e inevitabili componenti spirituali e la difficoltà, l'angoscia, la paura, le persecuzione e, soprattutto, l'impossibilità probatoria di dimostrare la relazione causale tra il fatto persecutorio e la condizione di assoggettamento, di angoscia e di pericolo nel quale la persona vittima si trova a operare. Quindi, abbiamo ritenuto che questa potesse costituire in un certo senso la porta per rimeditare un diritto di polizia, che si è abbandonato a suo tempo quando la giurisdizionalizzazione sembrava una soluzione inevitabile, ma al quale forse occorrerebbe ripensare se ci si convince che, per determinati delitti - e qui parlo del femminicidio - ciò che effettivamente può pagare la richiesta di giustizia della società è la prevenzione e non certo il diritto penale, che interviene quando un evento o la morte si sono già verificati. Signor Presidente, interrompo qui il mio intervento: dovrei parlare di svariati argomenti dei quali nessuno ha parlato, ma non è possibile farlo. Lo dico con grande sofferenza, perché di questo testo così complesso si è discusso soltanto dei reati contro la pubblica amministrazione: è davvero un aspetto che ci preoccupa, perché è dimostrativo del fatto che si ragiona sul nulla, su cose oltre tutto sulle quali siamo perfettamente concordi, auspichiamo che la Camera ponga la parola fine a una vicenda che a noi non è mai piaciuta, tant'è che in Commissione questo dibattito era evidente ben prima che gli altri ne parlassero. Nell'esprimere la mia personale adesione a un testo così significativo, complesso e dibattuto, devo comunicare all'Assemblea, che il Gruppo al quale appartengo ha deliberato di lasciare libertà di voto ai suoi componenti, che quindi decideranno di comportarsi secondo la loro personale coscienza.

27 e 28 giugno in Italia c'è stato un afflusso straordinario di migranti dal Mediterraneo centrale:

10.000 persone in più che hanno fatto arrivare la cifra complessiva dei migranti giunti nel nostro Paese dal gennaio 2017 a 85.000:

Mi sia consentito in quest'Aula - penso interpretando il sentire di tutti i Gruppi parlamentari - di ringraziare tutti coloro che hanno operato per affrontare questa straordinaria situazione: le forze di polizia, la Guardia costiera, la Marina militare, i prefetti, i sindaci, la Croce Rossa, i volontari. La situazione è molto difficile e impegnativa, ben sintetizzata dalle parole impegnate e impegnative del Presidente della Repubblica, in quel momento in missione internazionale. Abbiamo reagito su due versanti: il primo è stato quello di risolvere il problema sul terreno dell'accoglienza e il secondo di mettere in campo un'iniziativa politica che segnalasse immediatamente la situazione molto difficile nella quale l'Italia si è trovata. Abbiamo assunto un'iniziativa che - a mia memoria - è senza precedenti. Abbiamo inviato l'ambasciatore a Bruxelles presso la Commissione europea, per dire con grande chiarezza che, di fronte a quello che stava avvenendo nel Mediterraneo centrale e poi in Italia, l'Europa doveva assumersi maggiori responsabilità. Nelle ore successive, abbiamo chiesto un incontro con i principali Ministri dell'interno dell'Europa (il francese e il tedesco), al quale ha partecipato anche il commissario europeo Avramopoulos.

tra i principali Paesi europei e la Commissione, che potesse consentire di far arrivare chiaro un messaggio al vertice che domani si terrà a Tallin.

passo, confermato poi dalla Commissione europea attraverso la predisposizione dell'*action plan*. plan*. Considero veramente importante che la Francia, la Germania e la Commissione abbiano in qualche modo avuto una convergenza su una serie di nostre proposte. La prima è quella di un codice di comportamento per le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale. Non si tratta di una iniziativa estemporanea del Governo. C'è stato un intenso lavoro parlamentare di varie Commissioni, tra cui la Commissione difesa del Senato, che si è pronunciata con un documento approvato all'unanimità. Ed io che conosco le dinamiche parlamentari so perfettamente quanto sia impegnativo e soprattutto quanto sia forte il messaggio di un documento approvato all'unanimità.

Tuttavia, dal lavoro parlamentare emerge con evidenza che vanno poste due grandi questioni. La prima questione è quella relativa tra le attività delle organizzazioni non governative, tra le numerose navi che agiscono nel Mediterraneo centrale, nelle acque costiere libiche, con la Guardia costiera libica. E quello è un punto cruciale, perché è del tutto evidente che nelle acque territoriali deve operare secondo il principio di piena responsabilità. Tra mille difficoltà e con tantissimi problemi, negli ultimi mesi la Guardia costiera ha operato 10.000 salvataggi in mare. E queste cose le dice non il Governo italiano, ma l'Organizzazione mondiale per le migrazioni, la quale proprio ieri, nel riconoscere gli sforzi e i passi in avanti fatti sul terreno dell'iniziativa di salvataggio in mare - *search and rescue* - ha anche detto che la Guardia costiera libica ha salvato dalla morte

che ci deve essere un'azione della Guardia costiera nelle acque territoriali e tutte le altre attività, ivi comprese quelle delle navi delle organizzazioni non governative, devono svolgersi fuori dalle acque territoriali. La seconda questione che sarà posta nel codice di regolamentazione riguarda il coordinamento con l'attività di polizia giudiziaria nei confronti dei trafficanti di esseri umani.

numerose navi civili, un Paese serio prende tutte le misure per coniugare la salvezza della vita con le esigenze della propria sicurezza e l'assoluta necessità di essere inflessibili nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. Allora, come voi comprenderete - lo capirete ancora meglio quando leggerò dei dati - ci troviamo di fronte a una questione non di piccolissimo conto. Nei primi sei mesi Nei primi sei mesi di quest'anno, di fronte a 85.000 persone salvate, i numeri sono i

una bella pagina di cooperazione tra Parlamento e Governo. Il Parlamento fa un'indagine e propone; il Governo si muove in sintonia e la presenta in Europa, diventando così quella una posizione europea. Spero che sia così anche oggi, in questo Parlamento. Se non così fosse mi taccio, un po' stupito, ma mi taccio. ma mi taccio. È importante che, accanto a questa misura, l'Unione europea abbia impegnato la Commissione

E la Libia è un Paese chiave in questa partita; lì si gioca una partita cruciale: il 97 per cento delle persone arrivate nei primi sei mesi

In Libia dobbiamo misurarci con la fragilità e l'instabilità del Paese, ed è tutto molto più difficile.

Combattere il traffico di esseri umani significa di fatto aiutare la stabilizzazione della Libia. Naturalmente non è solo questo il problema - ci sono altre questioni che riguardano iniziative di carattere internazionale e diplomatico - ma è uno dei punti,

Il suo primo caposaldo, il controllo delle acque territoriali libiche, passa attraverso il rafforzamento, l'addestramento l'accresciuta capacità d'iniziativa della Guardia costiera. Abbiamo formato gli equipaggi nei mesi scorsi; abbiamo consegnato quattro motovedette alla Guardia costiera libica e altre ne consegneremo nelle prossime settimane e mesi. Nei Nei prossimi giorni, andrà a Tripoli per supporto logistico un pattugliatore della Guardia di finanza.

di finanziare e costruire - cosa che dev'essere fatta al più presto - un centro di coordinamento del soccorso marittimo a Tripoli. L'obiettivo è farlo entro la fine dell'anno, al massimo entro l'inizio dell'anno prossimo. Un centro di coordinamento per l'attività di soccorso a Tripoli costituisce un elemento importante, perché in questo momento, nel Mediterraneo centrale, agisce soltanto il centro di coordinamento e soccorso marittimo italiano. Avere un centro di soccorso marittimo a Tripoli, che quindi consenta alla Guardia costiera di poter operare nelle acque territoriali e, contemporaneamente, di riportare in Libia le persone che vengono salvate nelle acque territoriali, è un punto cruciale. Il secondo caposaldo è il seguente: poiché l'obiettivo è avere una Guardia costiera che controlli i flussi che partono dalla costa settentrionale della Libia per riportarli in Libia, è fondamentale

il rispetto dei diritti umani, e su questo io penso che il Parlamento italiano non possa che essere profondamente intransigente.

l'UNHCR, che gestisce dette questioni per le Nazioni Unite, è andata per la prima volta a Tripoli. Ora, naturalmente si tratta di implementare tutto questo lavoro. Si tratta di trovare un più forte e significativo sostegno e il fatto che l'Europa investa di più al riguardo - voi comprendete - significa affrontare un altro piccolo tassello

Il confine Sud della Libia è il confine Sud del Mediterraneo centrale e, quindi, è il confine Sud dell'Europa. Non è il confine Sud dell'Italia. Se qualcuno pensa che il Sub-Sahara sia il confine Sud dell'Italia, fa un drammatico errore. Il Sub-Sahara è il confine dell'Europa. Sulla sua sicurezza si gioca una partita fondamentale per il futuro dell'intero continente europeo. Nelle settimane scorse sono venute a Roma le tribù principali, i cosiddetti guardiani del deserto - i Tebu, i Tuareg, i Suleiman - che erano in guerra tra di loro e hanno firmato la pace di fronte al Governo italiano. l'hanno fatto al Ministero dell'interno, al Viminale, esprimendo una fiducia molto forte nei confronti del rapporto con il nostro Paese. Quelle tribù potranno costituire, domani, la spina dorsale di una moderna guardia di frontiera libica per tutelare i confini meridionali della Libia, insieme con altri due Paesi chiave con i quali abbiamo chiuso un accordo di cooperazione, il Niger e il Ciad. Voi comprendete, quindi, che incomincia a vedersi una prospettiva di intervento organico dall'altra parte del Mediterraneo. Nei prossimi giorni andrò a Tripoli per incontrare i sindaci libici e discutere con loro di progetti concreti di sviluppo e cooperazione. Nel momento in cui ci poniamo l'obiettivo di stroncare il traffico di esseri umani - cosa assolutamente indispensabile e immediata, perché si tratta di una guerra senza quartiere e poiché in questo momento il traffico di esseri umani è forse l'unica industria che funziona in Libia, forse l'unica realtà che produce, in modo criminale e nella maniera più distorta possibile, una redistribuzione del reddito

Il consenso delle comunità locali è fondamentale nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, per l'accoglienza in Libia e nella lotta contro il terrorismo. Il 24 luglio a Tunisi faremo la seconda riunione - la prima si è fatta a Roma - del gruppo di contatto tra Europa e Africa settentrionale. Sarà un momento importante per fare il bilancio di questa complessa strategia. La Commissione europea ha messo a bilancio 153 milioni per quest'anno e 200 milioni per l'anno prossimo, ma non non bastano. C'è bisogno di un impegno diretto dal punto di vista finanziario dei singoli Stati membri. C'è una sproporzione evidente tra quello che si è investito sulla rotta balcanica e quello che si sta investendo nel Mediterraneo centrale. Per me non è comprensibile e accettabile. È importante che vi sia una strategia comune dell'Europa sui rimpatri. I rimpatri sono un punto cruciale e fondamentale per ogni politica di immigrazione. In questo momento l'Italia ha prodotto un più 26 per cento per quanto riguarda gli allontanati e un più 16 per cento per quanto riguarda i rimpatri.

decide di adottare una strategia comune per quanto riguarda i rimpatri, accoglie una richiesta storica che l'Italia ha sempre avanzato. Soprattutto c'è un'altra questione: accanto ai rimpatri l'Europa è disponibile - vedremo domani a Tallin - ad applicare una politica comune dei visti.

Noi abbiamo flussi notevoli e significativi da Paesi che vengono considerati assolutamente sicuri. Le persone che vengono da Paesi sicuri vanno rimpatriate. C'è bisogno di accordi di riammissione e di disponibilità nella riammissione. Se un Paese

comunicare la loro intenzione di aumentare le *relocation* verso i propri Paesi non lo considero assolutamente risolutivo, ma è un piccolo passo in avanti.

Tuttavia, in questi giorni si è posta un'altra questione di assoluto rilievo, che è giusto affrontare apertamente in Parlamento. ultimi anni l'Italia ha dato una straordinaria prova di accoglienza: lo ha fatto, lo sta facendo e lo farà. L'accoglienza è scritta nel DNA del popolo italiano e del Paese. Tuttavia, mi chiedo e vi chiedo si può separare la salvezza in mare dalla terra che accoglie. Se non ci sono la terra e l'approdo, la salvezza è soltanto provvisoria. Separare la salvezza e l'accoglienza rischia di apparire una gigantesca ipocrisia. ipocrisia. È difficile pensare che ci possano essere una missione internazionale di salvataggio e un solo Paese che accoglie le persone che sono salvate: questo è il cuore della questione che abbiamo posto.

Ho la sensazione che, in questo caso, una parola modernissima come questa non funzioni. Temo che si tratti di tornare a qualcosa di più antico, che è sempre stato nelle vene dell'Europa tutta, ma soprattutto nelle vene dell'Europa mitteleuropea. La parola è questa: etica della responsabilità. L'Europa che non comprende questo è un' Europa che rischia di perdere se stessa.

di inviare una lettera a Frontex, per chiedere un'immediata e urgente riunione, per ridefinire le regole della missione Triton, affrontando il tema della regionalizzazione dei soccorsi, con pazienza, con capacità di ascolto delle ragioni altrui, e con la fortissima convinzione delle nostre ragioni, così come abbiamo fatto ieri, quando a un certo punto è apparso sulle agenzie di stampa che il Ministro della difesa austriaco aveva minacciato di schierare truppe ai confini con il nostro Paese. Di fronte a quelle dichiarazioni abbiamo risposto dicendo fondamentalmente tre cose. La prima è che non c'era alcuna emergenza al Brennero. La seconda è che la cooperazione tra le forze di polizia italo-austriache era ottima. La terza è che Italia e Austria avevano una lunga tradizione di amicizia e di cooperazione. Oggi è intervenuto su questi temi il cancelliere della Repubblica austriaca, il quale ha detto sostanzialmente tre cose: non c'è alcuna emergenza al Brennero; tra Italia e Austria c'è una straordinaria cooperazione tra le forze di polizia; i rapporti tra Italia e Austria sono sempre stati improntati ad amicizia e cooperazione. Prendo atto. Noto pacatamente che forse avevamo ragione noi. Con Con questo spirito andiamo domani a Tallin al vertice informale dei Ministri dell'interno dell'Unione europea. Con questo spirito affronteremo la discussione nei prossimi giorni in sede Frontex. Mi avvio alla conclusione. Abbiamo di fronte una vicenda epocale, incominciata molti anni fa, quando forse fu commesso il vero peccato originale di questa situazione, e cioè il Trattato di Dublino del 2003. È una vicenda incominciata molti anni fa che probabilmente accompagnerà il mondo, non l'Italia, per ancora altri anni. Un grande Paese come l'Italia non subisce, non insegue. Un grande Paese come l'Italia deve avere l'ambizione di governare questi processi, che sono connaturati, un pezzo della storia del mondo, e non soltanto di una parte di questo mondo. Se qualcuno avesse qualche dubbio, basta sollevare un attimo lo sguardo dai nostri problemi e guardare quello che avviene nel pianeta per capire cosa significano queste parole. Se questo è il tema, non ci sono formule magiche; bisogna parlare un linguaggio di verità al Paese; non ci sono semplificazioni rafforzate. Ci vogliono una visione organica, una strategia, un impegnativo e un impegnato lavoro di costruzione. Vedete, illusione è una parola straordinariamente bella. L'illusione si afferma velocemente, ma poi, altrettanto velocemente, può rovesciarsi nel suo opposto, la disillusione. Attenti, e lo dico innanzitutto a me stesso: l'onda della disillusione è molto più forte del soffice vento dell'illusione. Ma per me, proprio perché dico questo, c'è un punto cruciale un punto cruciale che è il seguente. Ho detto più volte, in varie sedi parlamentari, che ritengo sbagliata l'equazione tra terrorismo e immigrazione. Tuttavia, se guardiamo l'Europa degli attacchi terroristici, da «Charlie Hebdo» in poi,

Se questo è il tema, bisogna dire con grande chiarezza - come io dico questa sera in Parlamento - che l'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione. Per quanto mi riguarda, è un limite invalicabile. Su questo mi sento personalmente impegnato: il Ministro dell'interno non può non comprendere che su questo si giocano il presente e il futuro del nostro Paese. La sicurezza è uno straordinario bene comune di tutti gli italiani. Ho concluso. Vi ho detto ciò che penso. Può piacere o meno; è la forza e insieme la bellezza della democrazia. Tuttavia, consentitemi di dirvi un'ultima cosa: su questi temi non si gioca soltanto la partita del consenso. In democrazia la partita del consenso è importante, ma non si gioca soltanto questa. Su questi temi si gioca qualcosa in più, la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese. Si gioca un pezzo del futuro della nostra democrazia. Se questa è la sfida, questo Parlamento, anche in vista degli appuntamenti internazionali dei prossimi giorni, ha più ragioni per unirsi e non per dividersi.

PLI))*. Signor Presidente, signor Ministro, mi consenta innanzitutto di associarmi al ringraziamento che lei ha formulato nei confronti delle nostre Forze armate e di quanti operano su un fronte così difficile.

la necessità che un grande Paese assicuri la salvezza della vita umana, ma anche la propria sicurezza, ragion per cui nessun grande Paese, per quanto grande, può accogliere illimitatamente flussi migratori. Ciò è ancora più importante perché per troppo tempo il nostro Paese non ha avuto un'iniziativa e la situazione che ci troviamo oggi di fronte è anche

costruendo grandi centri che potessero produrre grandi indotti sia economici che politici, allungando i tempi di esercizio delle commissioni e attendendo che una parte di quanti arrivavano nel nostro Paese andassero via. Questa non è una politica e io riconosco che, rispetto a questo passato prossimo, c'è una differenza. Signor

Il suo collega e predecessore, il ministro Alfano, pochi giorni fa, in un incontro con il Qatar, ha detto che il problema non è la Libia.

e dovremmo anche ammettere che la nostra posizione in Libia non è chiara. Abbiamo puntato su Serraj, un'autorità a a termine, e ci troviamo in una situazione nella quale il Paese è fuori controllo, diviso tra Haftar da una parte e Fratelli musulmani dall'altra. Tale divisione ci ricorda molto quella che esiste tra sauditi ed egiziani da una parte e Qatar dall'altra, ma non si sa da quale parte stiamo noi. Non si sa quale sia la nostra strategia per arrivare alla stabilizzazione di quel Paese che lei ci ha detto essere essenziale per risolvere il problema. Possiamo chiedere al Governo con chi stiamo? Possiamo chiedere se è arrivato il tempo di mettere fine a una politica diplomatica nei confronti dell'Egitto assolutamente irresponsabile? Altro che etica della responsabilità! Siamo ancora senza un ambasciatore al Cairo. Signor Ministro, lei ha impostato un programma nel quale, a quanto ci ha detto, i segnali politici sono molto importanti.

a quelle navi che battono bandiere di altri Paesi (saranno una minoranza, ma ci sono) di entrare nei porti di quei Paesi, anziché dare ospitalità. Perché questo non è possibile? È un segnale che farebbe capire che quella etica della responsabilità alla quale lei ha fatto riferimento deve essere una etica della responsabilità di tutti, non una etica di responsabilità che vale solo per il nostro Paese.

che è mio possa essere anche suo. Ma le sembra un segnale, in una situazione del genere, accingerci all'approvazione di una legge come lo *ius soli*, che delega ad altri un diritto personalissimo come quello della cittadinanza, che lei, come me, sa poter essere esercitato soltanto dopo il diciottesimo anno di età? Per quale motivo delegarlo ad altri, fossero anche i parenti più prossimi, nel momento in cui lei ha fatto riferimento ai rischi di una mancanza di integrazione e a quanti problemi abbia causato nel resto d'Europa il fatto che vi sono stati giovani che non hanno scelto la loro cittadinanza ma se la sono trovata derivata, e abbiamo avuto il terrorismo legato all'immigrazione di seconda o terza generazione? Signor Ministro, io spero che il Parlamento possa produrre una risposta unitaria. Ma allora questi dubbi non devono essere soltanto i dubbi di una parte, ma i dubbi di tutto l'emiciclo. Presidente, ministro Minniti, sono almeno quattro anni che state cercando di far credere al Paese che in tema di gestione dei flussi migratori la politica italiana riesce a condizionare quella europea. È falso! Sulla chiusura dei porti italiani per gli sbarchi avete già subito un secco no da Spagna e Francia, da quel Macron che avrebbe contribuito alla piena intesa di Parigi con la Merkel, che poi è saltata. Da quel Macron che vi ha ricordato che l'80 per cento dei migranti che noi accogliamo sono economici, dunque clandestini, come la Lega dice da sempre! A Tallin discuterete di un piano d'azione frutto di alcune conclusioni dell'indagine sulle ONG fatta in Senato, realizzata dopo che la Lega Nord a febbraio ha chiamato il procuratore Zuccaro in Comitato Schengen, da dove è partito tutto. Se non fosse stato per noi è probabile che di ONG e di aree SAR in Parlamento non se ne sarebbe parlato ancora a lungo. E anche il Movimento 5 Stelle non avrebbe virato la propria rotta di 180 gradi sulla politica dell'immigrazione. Discuterete a Tallinn di centro di coordinamento in Libia (ci vorranno mesi, se non anni), di creazione di aree di salvataggio in Tunisia e in Libia, di codici di condotta per le ONG. Porterà a casa qualche altro milioncino, dimenticando che noi spendiamo quest'anno quasi cinque miliardi di euro. Ma le domando: perché su Malta nessuna pressione per rimediare finalmente al loro mancato recepimento della direttiva IMO in materia di porto sicuro? È l'unico Paese europeo a non avervi proceduto, eppure Malta, fino a poche ore fa, Presidenza del semestre europeo. Così noi continueremo ad essere l'unico porto sicuro del Mediterraneo. Dal vertice per l'ennesima volta il Governo porterà a casa poco, come avvenuto nei Consigli europei degli ultimi tre anni; come è accaduto con i tre pilastri fissati nei Consigli europei del 2015. Ricordo ancora Alfano che, tronfio, parlava di *hotspot*, rimpatri e ricollocamento. Gli *hotspot* li abbiamo subiti; sui rimpatri c'è stato un fallimento, perché avete azzerato il Fondo rimpatri; è fallito anche il ricollocamento, ma qui le cause che voi attribuite all'egoismo di alcuni Paesi dell'Europa in realtà erano chiare da subito e la Lega vi aveva avvertito.

Eppure voi, per giustificare i vostri fallimenti, siete sempre alla ricerca di un capro espiatorio: l'Europa o la comunità internazionale. Da loro non otterrete risultati; magari da taluni Paesi per egoismo, ma soprattutto perché la gran parte non si fida dell'Italia per la sua politica permissiva, senza rigore, senza deterrenza, ammalata di buonismo e dunque di ipocrisia. da lei proposto si è persa un'occasione, ma comprendiamo: lei è prigioniero della sua stessa maggioranza. Si poteva e doveva, ad esempio, eliminare la protezione umanitaria (siamo l'unico Paese a riconoscerla); aumentare il Fondo rimpatri; potenziare le operazioni di rintraccio di immigrati irregolari nel nostro Paese: tutte proposte della Lega che sono state bocciate. In compenso, la maggioranza ha approvato ancora l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina; ha detto di sì ad un gravissimo ordine del giorno che prevede la riduzione del ricorso all'allontanamento dei migranti. Questa è la verità. In Italia ci sono troppi fattori di attrazione che voi, nel tempo, avete irresponsabilmente accresciuto, e che attraggono migranti economici, dunque clandestini. ancora il sistema di accoglienza, che elargisce servizi per tutti, quando abbiamo 7,7 milioni di italiani in stato di deprivazione. Ci sono tempi lunghi per l'esame delle richieste d'asilo pochi rimpatri; ci sono poi gli interessi economici di cooperative e private, ma anche della criminalità organizzata, che vogliono alimentarsi con l'industria dell'accoglienza. Ci sono le ONG, ma c'è soprattutto la volontà politica: una maggioranza trasversale in Parlamento *pro* immigrazione, che punta all'accoglienza a tutti e a tutti i costi. Ministro Minniti, vada a Tallinn e tratti di questioni con l'Europa e con la comunità internazionale ma - si ricordi - faccia subito azioni di politica interna; lavori per diminuire i fattori i fattori di attrazione del nostro Paese; attui rigore e legalità. Più rintracci; più controlli alle frontiere terrestri; più riammissioni attive, non subisca solo quelle passive; più rimpatri; più capienza nei centri di permanenza per il rimpatrio. Aumenti i tempi di trattenimento, come previsto dalla direttiva sui rimpatri; non ammetta richieste d'asilo per manifesta infondatezza per coloro che vengono da Paesi sicuri. Signor Ministro, applichi queste proposte; diversamente proseguirà ancora di più l'invasione; diminuisca i fattori di attrazione interni per governare e ridurre l'immigrazione clandestina: questa è un'immigrazione incontrollata che non va bene, che va a scapito non solo degli italiani, ma anche degli extracomunitari regolari e dei pochi rifugiati. Signor Ministro, diminuisca i fattori di attrazione. Invece, la sua maggioranza e il suo Governo cosa fanno?

che è fuori controllo e sta creando problemi pazzeschi al Paese e alle comunità locali. I dati mancano da due mesi e mezzo e nel cruscotto giornaliero sul sito del suo Ministero i dati che si estrapolano, ancorché vecchi, dicono che mancano 50.000 presenze. Dove sono tali presenze? Risponda alle nostre interrogazioni parlamentari; riporti un po' di trasparenza, che sta sempre più venendo meno. Non lo deve a noi del Gruppo Lega Nord, ma lo deve deve soprattutto agli italiani. Signor Ministro, mi complimento con lei personalmente perché è sicuramente persona

di ben 123.000 profughi, cioè circa 10.000 ogni mese. Solo nel triennio 2014-2016 l'Italia ha accolto sulle proprie coste circa 500.000 migranti, più di quanti ne sono arrivati negli ultimi

Per quanto riguarda la nazionalità, sappiamo che arrivano soprattutto dal Nord Africa (Nigeria, Senegal, Gambia, Eritrea). A questo punto, non crediamo si possa più definire semplicemente emergenza un fenomeno che, ahimè, sta diventando stabile. Non possiamo più, quindi, fronteggiare questi problemi, che sono strutturali, con risposte valide solo per meccanismi emergenziali. Ciò significa che non possiamo porci solamente le domande di quanti migranti arriveranno e di quanti ne dobbiamo nutrire Certo, sono domande a cui bisogna dare risposte nell'emergenza, ma non basta. Si deve andare oltre, bisogna fare la diagnosi precisa per fare una terapia adeguata.

poveri cristi che fuggono da Paesi politicamente instabili; fuggono dalle dittature, da situazioni gravi, spesso da guerre e persecuzioni. Questi soggetti vanno verso l'Europa inseguendo un miraggio, una luce. L'Unione europea è chiaramente in difficoltà rispetto a questo problema e, del resto, siamo forse stati un po' superficiali.

la grande questione sociale del nostro tempo consiste nell'enorme divario tra il Nord e il Sud del mondo. Qui - nel Sud - sono iniziate correnti migratorie che, in assenza di un processo di sviluppo che abbracci tutta la riva del Sud del Mediterraneo, sono destinate a gonfiarsi in maniera impressionante e saranno

possibilità di sviluppo, certezze. Tutto ciò nasce quindi dalla frustrazione, dall'insufficienza e dalla cattiva costruzione di rapporti sulla base del colonialismo e del *post*-colonialismo dei Paesi occidentali. La mia diagnosi detta in soldoni, caro Ministro, è questa: lì c'è uno stato di bisogno, c'è la guerra, c'è tutto il male del mondo; tenta di andare via e a questi bisogni risponde la criminalità che si organizza per fare *business*, per fare guadagno - soprattutto la Libia - e li porta da noi.

intervenendo anche sul tema dell'integrazione. Auspichiamo quindi, signor Ministro, che domani a Tallin, si possa parlare concretamente non solo di fondi e di impegni contingenti dei Paesi europei, ma anche di soluzioni radicali, di visioni strategiche,

le vorrei ricordare che non solo il Regno delle due Sicilie già controllava il Mediterraneo e le coste del Nord Africa, ma prima ancora le controllava

Dobbiamo costringere l'Unione europea e la comunità internazionale ad intervenire con noi e se non lo fanno lo faremo da soli. Così si diventa uno Stato autorevole. Lo faremo da soli anche a costo di ritirare la nostra partecipazione economica alla Comunità europea.

che chiama in causa le politiche di sviluppo dell'Occidente degli ultimi vent'anni e le responsabilità - italiane e comunitarie - verso un fenomeno migratorio di portata globale. Di fronte a questi elementi, sarebbe fondamentale una visione nazionale e condivisa, chiara e di ampio respiro. Ci troviamo di fronte ad uno dei grandi temi della storia di questo secolo: accettiamo la sfida, accogliendo la possibilità di essere impopolari nei sondaggi ma giusti nei confronti di un'umanità che che fugge da guerre, desertificazione, povertà. Una caustica vignetta di Altan di qualche giorno fa aveva questa didascalia: «Che cosa sono i migranti economici? Quelli che hanno paura di morire di fame invece che per le bombe». Certo, migrare non è un diritto, ma non è nemmeno immaginabile chiudere la porta in faccia a chi cerca un luogo dove poter sopravvivere dignitosamente. Per troppi anni il Continente africano è stato trattato come una riserva senza fondo dai Paesi del cosiddetto "Primo mondo". Abbiamo distrutto ed inquinato i suoli per l'estrazione di petrolio, minerali e diamanti, sfruttato i lavoratori, e flotte di pescherecci con reti a strascico davanti alle coste senegalesi lasciano ben poche possibilità ai pescatori locali che usano piccole barche di legno per sfruttare le risorse del mare. Questo è solo un esempio, così come nei prossimi anni sempre più persone saranno costrette ad abbandonare le loro terre per gli effetti dei cambiamenti climatici. Tuttavia, la complessità del problema andrebbe quindi affrontata con parsimonia parsimonia di dichiarazioni improvvisate. Al contrario, in troppi contribuiscono a creare rumore di sottofondo. Lo stigma è oggi nei confronti delle ONG, ree di essere fattore di attrazione, circostanza ampiamente smentita dai dati più recenti È utile rammentare che a fine 2013 il Governo italiano aveva intrapreso coraggiosamente la missione Mare nostrum per svolgere le operazioni di soccorso in mare. In quel contesto era possibile avere le nostre forze di polizia a bordo delle navi della Marina militare, con un presidio sanitario efficiente. Come ben sappiamo, Mare nostrum è stata sostituita da altre operazioni, creando le condizioni per lo sviluppo del presidio in mare da parte di organizzazioni non governative provenienti da vari Paesi. Parliamoci chiaro: abbiamo affrontato questa tematica in modo scomposto ed estemporaneo, dando alla Commissione difesa il compito di produrre una strategia che contemperasse la presenza delle ONG con quella delle forze in mare. Non poteva che uscirne una proposta frammentaria, come la richiesta di collocare operatori di polizia giudiziaria a bordo delle navi battenti bandiera straniera. Mi resta la curiosità di capire con quale autorità possiamo pretendere di avere ufficiali di polizia giudiziaria su suolo straniero, perché di questo stiamo parlando quando ci riferiamo a navi straniere in acque internazionali. internazionale (ISPI) ha evidenziato che, al 27 giugno di quest'anno, sono stati ricollocati in Europa solo 7.277 richiedenti asilo di quelli arrivati in Italia. Questo confligge con l'impegno dell'Europa assunto nel 2015, il quale prevedeva la ricollocazione di circa 35.000 richiedenti asilo verso altri Stati membri entro settembre 2017. Anche se l'Unione europea avesse mantenuto fede all'impegno sui ricollocamenti, avrebbe sollevato l'Italia solo per il 10 per cento del totale delle richieste d'asilo dal 2013 a oggi. Non limitiamoci però soltanto ai dati, ma proviamo a pensare anche alle potenzialità che abbiamo per risolvere il problema. Chi, come il sottoscritto, ha avuto modo di visitare il Comando in capo della Squadra navale (Cincnav) sa bene quale siano le capacità militari e di sorveglianza impiegate. Pertanto, un eventuale posizionamento delle navi militari meno lontano dal limite delle acque territoriali libiche riuscirebbe a garantire un controllo maggiore su cosa avviene nelle operazioni SAR, potendo così evitare che scafisti armati continuino ad agire quasi indisturbati.

La Libia è uno Stato polverizzato, un Paese con 1.700 chilometri di coste e oltre 4.000 chilometri di confine su terra, con Algeria, Chad, Egitto, Niger, Sudan e Tunisia. Nessuno di questi Paesi confinanti è sicuro, ma sono confortato dall'impegno del Governo attraverso programmi di cooperazione allo sviluppo. infine, che per il 2017 l'Italia è anche membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una posizione dalla quale far sentire con maggior forza la nostra voce per chiedere un impegno globale sui migranti, ma soprattutto la costruzione di corridoi umanitari per per affrontare il dramma dei rifugiati nelle regioni più a rischio e per la lotta ai trafficanti di esseri umani, che fanno affari con chi fugge dalle guerre e carestie. Il prossimo novembre avremo anche la Presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e credo che quella sarà l'occasione giusta per porre il problema.

Lei è capacissimo, persona che conosce e sa, però dobbiamo renderci conto che mentre il medico studia,

non saremo in grado di controllare quello che accade in un Paese che sta attraversando anche una crisi più generale. E allora qualcosa di concreto per frenare quest'ondata anomala e incredibile verso l'Italia va fatto. Non illudiamoci che lo farà qualcun altro con noi, signor Ministro: lo stanno dimostrando e l'hanno già dimostrato quando si è voluto intervenire per le primavere arabe; i «sì» francesi e inglesi dove stanno adesso

Ha dell'incredibile tutto questo: alla faccia della solidarietà! Sia ben chiaro, sono favorevole all'Europa, ma mi rendo conto che siamo soli. siamo soli. Si è commesso un errore quando si è fatto l'accordo con la Turchia, tutto si è bloccato e non si è pensato a questa parte. Lì il problema non c'è più e gli egoismi li abbiamo tutti sull'Est Europa, che non ci verrà incontro, nonostante gli enormi sforzi che lei compirà a Tallinn domani. Me ne rendo conto, ma la Germania e la Francia devono essere più chiare e più vere. L'Italia non può diventare il Paese in cui vengono a fare *shopping*, anche economico e finanziario, perché possono pensare di tutto nel metterci in crisi. Non ci bastano 100 o 200 milioni,

abbiamo la seconda o terza generazione di terroristi. Su questo dobbiamo ragionare tutti e a tutti vorrei dire che questi problemi non si affrontano con le ideologie o con le convinzioni di provenienza. Il problema è reale e concreto e va affrontato dall'Italia seriamente.

altri soccorrono: queste ONG viaggiano, fanno, prendono e arrivano nei porti italiani. Chi sono? Perché? È mai possibile che non si possa raccordare tutto questo? È mai possibile che non possiamo controllare tutto questo, noi che siamo vittime del problema? Nessuno può accusare il popolo italiano di non avere carità cristiana e accoglienza. Ne abbiamo sempre date e avute siamo pronti a darne, ma non possono chiedere al popolo italiano di morire, perché ha già problemi propri, per queste situazioni abnormi che sembrano non interessare assolutamente all'Europa. Anche adesso ne avete avuto i risultati: siamo alle parole,

non inteso nel senso destroide o altro - le chiedo che l'Italia alzi la voce. Siamo stati sempre il Paese della disponibilità e del dialogo, veniamo da una cultura di questo tipo. Oggi è il momento in cui Francia e Germania capiscano che l'Italia si è seccata, ha dato e vuole dare, ma vuole rispetto: se gli altri non ce lo danno, non lo potranno riceverlo da noi. Un nostro indebolimento favorirà altre politiche economico-finanziarie di francesi e tedeschi sul nostro territorio e lei sa che questo avviene. Di questa gente diffido,

dal nostro impero sono venuti somali ed etiopi e li abbiamo accolti. Quanti etiopi, somali o eritrei sono in Italia e sono medici? Ma non era un problema, era un problema, se non da gestire. Oggi non è così, è quasi un'invasione di ogni tipo e specie, che può portare guai seri, e li sta portando. La mia preoccupazione è la coesione sociale del Paese, che è già indebolito da problemi economici. Ministro, occorre un'azione più concreta e reale: a lei non mancano né la preparazione, né la competenza, né la forza per affermare questo. Credo che se l'Italia

serve solo a questo perché mi rendo conto che nei momenti importanti bisogna essere uniti. Certo, resta lo sgomento di vedere quest'Aula quasi deserta.

di *partner* dell'Unione europea, che alcuni Stati si sottraggano alle loro responsabilità, voltando le spalle e lasciando sola l'Italia ad essere frontiera dell'Europa. Se noi ci assumiamo delle responsabilità, a queste responsabilità gli altri Paesi, in particolare la Francia, la Spagna anche l'Austria, non si possono sottrarre. In altri termini, ogni chiusura unilaterale di fronte alle esigenze di coordinamento, di condivisione e di controllo comune, è destinata ad avere una grave conseguenza sull'Unione europea stessa. I problemi possono essere risolti esclusivamente insieme, solo assieme si governano i flussi migratori, i maggiori e più efficaci controlli delle frontiere esterne e delle frontiere meridionali della Libia, l'introduzione di un codice di condotta per le ONG nel Mediterraneo, il rafforzamento delle misure sui rimpatri e, nel contempo, la riallocazione dei migranti presenti sul territorio degli Stati europei. Come ha ribadito il Governo italiano, tale condivisione è indispensabile e se tale condivisione non c'è, allora anche l'Italia sarà costretta a prendere misure unilaterali, forse anche estreme come il blocco dei porti, ma speriamo che non si arrivi Voglio aggiungere questo: le azioni che sono state minacciate alla frontiera del Brennero, ossia di schierare l'esercito e i mezzi blindati, sono assolutamente ingiustificate. è spazio per queste misure e per questi comportamenti manifesto, che non sono giustificati nemmeno in vista delle elezioni politiche. Sono inutili e dannosi anche per il clima di ottima collaborazione che c'è tra l'Italia e l'Austria proprio per il controllo dei flussi migratori. I risultati sono di tutta evidenza: i flussi migratori dall'Italia verso l'Austria non sono affatto aumentati la situazione è perfettamente sotto controllo anche grazie all'impegno dei ministri dell'interno, prima Alfano e oggi Minniti. Bisogna anche aggiungere che, allo stato, il numero dei migranti che rientrano dall'Austria verso l'Italia è lievemente superiore a quello che va nella direzione opposta

Restiamo quindi convinti come ogni ulteriore errore e il perdurare dell'inerzia diminuiscano la capacità dell'Europa di essere un soggetto geopolitico unitario. Ciò renderebbe meno credibile e meno forte in primo luogo il piano di azione proposto dalla Commissione europea stessa e insostenibili i flussi migratori. Dobbiamo quindi operare per una svolta, come ha detto anche il ministro Minniti, nel sud del Mediterraneo, anche con la creazione di aree di soccorso e di permanenza in Libia e in Tunisia. Il Centro unico di comando europeo proposto dall'Italia rimane una proposta che consideriamo fondamentale che il Governo, giustamente, continua a

che il Governo che sosteniamo ha le idee chiare su questo punto. Il Ministro ha detto anche un'altra cosa. Francamente questo pomeriggio, venendo ad ascoltare l'amico ministro Minniti, avevo un timore. Vi confesso che la mia fede ha vacillato, perché ho temuto che Minniti venisse qua a spiegarci i risultati (sarebbe stato anche umano se lo avesse fatto) della sua azione diplomatica presso gli altri Ministri. Non ha ceduto a questa tentazione, perché ha parlato di «piccoli passi» nella direzione giusta (perché è chiaro che in questa circostanza ci mancherebbe altro che i piccoli passi fossero andati in un'altra direzione). piccoli passi e mi fa piacere anche questa prova di realismo. Non c'è trionfalismo, non poteva esserci e guai se ci fosse stato. Colleghi, la realtà delle cose è molto chiara: abbiamo la Spagna che ha davanti a sé due Paesi, come il Marocco e l'Algeria, che fanno un controllo sulle partenze, nel senso che da lì non si parte o si parte in misura limitata. Abbiamo un Paese come la Germania, che quando si è aperto un rubinetto dalla Turchia, ha avuto un'interlocuzione con il governo Erdogan, che possiamo criticare ma certamente dobbiamo riconoscere che esiste ed è forte. Quel Governo è stato in condizione di chiudere quei rubinetti. Poi abbiamo la Francia che pensa a tappare bene a Ventimiglia i buchi possibili, nonostante le professioni europee - che ho apprezzato - di Macron in campagna elettorale, che aspettiamo di vederle tradotte nei fatti. E l'Italia davanti chi ha? un non-Stato, a causa di un'azione dissennata che è stata fatta e che abbiamo pagato noi. E chi ha compiuto quell'azione non ha nemmeno sostenuto il Governo che l'ONU ha insediato, perché è andato a flirtare con Haftar. Ci troviamo quindi in una condizione per cui siamo disarmati,

tutto quello che è lo sforzo che chiediamo si limiterà a qualche soldo in più da dare alla Libia o ai Paesi dell'Africa subsahariana un piano B lo dovremo coltivare. Non credo che, agli effetti del diritto internazionale, sia ammissibile un blocco dei porti, ma

la possibilità di essere intercettato. Dunque, perché lì chiudono? Perché evidentemente hanno un collegamento con i trafficanti, come in fondo i magistrati hanno denunciato nella encomiabile indagine, che ha condotto il nostro collega e amico senatore il piano B deve consistere in qualcosa. Se una ONG batte bandiera spagnola, vada a scaricarli alle Baleari o, se batte bandiera francese, vada in Corsica. Oppure, ci può essere qualcos'altro,

ma importanti, che sarebbero stati fatti nell'ultima settimana. Per carità, ha fatto bene a chiedere un pre-vertice, ma purtroppo le cose non sono andate esattamente come le ha descritte. Ha assicurato che l'Europa si sta avviando verso quella condivisione di responsabilità invocata dall'Italia, ma cercare di addolcire la pillola, negando la realtà, non è mai una buona idea. Ciò aiuta forse nell'immediato, a a presentare all'opinione pubblica una situazione migliore, ma a nostro avviso è una strategia dal respiro corto, che finisce puntualmente per peggiorare la situazione. Conviene essere onesti, signor Ministro, e ammettere che, sul fronte dell'Unione europea, la pillola è amarissima.

La Francia del nuovo presidente Macron, è stata tra i principali responsabili del disastro libico, cui ci siamo accodati, anche se sento dire in quest'Aula che non si sa chi è stato a bombardare la Libia.

La Francia ha risposto riaffermando piena indisponibilità, la Spagna è stata un po' più garbata nei modi, ma non nella sostanza, e l'Austria, dopo le proteste dell'Italia, ha parlato oggi di equivoco e ha assicurato che i suoi carri armati resteranno nelle caserme, se i flussi migratori non aumenteranno. Non c'era bisogno di dire di più: il segnale è stato comunque inequivocabile. Nel piano della Commissione europea ci sono quelli che a Roma, la mia città, vengono chiamati "pannicelli caldi": uno stanziamento che sarebbe esagerato definire congruo. Lei lo sa perfettamente, signor Ministro: non c'è nessuna vera pressione per forzare la mano ai tanti Paesi europei, che non intendono assumersi alcuna responsabilità. Altro che etica della responsabilità! Sullo sfondo c'è solo la promessa,

che si sarebbe già dovuto fare da tempo, perché è l'unico che ci permetterebbe di affrontare in maniera più adeguata e di fronteggiare meglio la situazione, ma che è reso impossibile soprattutto dal veto dei Paesi dell'Est. Di fronte a questo ennesimo fallimento politico, alla fine l'Europa e l'Italia non hanno trovato - e mi spiace

La decisione è stata quella di coprire il solito nulla di fatto, con una stretta su chi in questi anni più di ogni altro si è adoperato per salvare vite umane. Non poteva però, me lo lasci dire, essere fatta una scelta più cinica. È bene chiarire che questa mossa decisa solo per nascondere l'insipienza dell'Europa

cose con il loro nome e non nascondere la realtà dietro formule anonime come «nuovo codice per le ONG». Del resto, basterebbe ascoltare chiunque si occupi davvero del soccorso ai migranti per fugare ogni eventuale dubbio su cosa comporteranno le nuove regole. Il senso politico di tutte queste scelte, che si cercano di presentare fragoroso sul piano mediatico, ma che sono inutili e spesso controproducenti su quello concreto, sarà evidente a breve. Di fronte alla pressione dei movimenti antieuropeisti, l'Unione e i singoli Paesi che ne fanno parte cercano di mettersi al riparo, assumendo come propri alcuni dei peggiori argomenti di quelle forze antieuropee. È una strategia che non funzionerà, da nessun punto di vista, perché cedere sul terreno dei valori e addirittura su quello della salvaguardia della vita non è un baluardo, è una resa. Il baluardo è invece mantenere, difendere e rafforzare i princìpi di solidarietà Significa creare corridoi umanitari, garantire protezione ai bambini, reclamare dall'Europa quell'assunzione collettiva di responsabilità che basterebbe a rendere del tutto tollerabile per tutti il flusso migratorio, attraverso l'etica di responsabilità che è tipica della cultura e della religione protestante. E guardi, proprio qui, in questo Paese, sono proprio la Tavola valdese e le Chiese evangeliche che stanno dando prova, con i corridoi umanitari che lei dovrebbe conoscere, di fare qualcosa di davvero funzionante e di concreto. Credo infine che bisogna stare molto attenti ai toni che si usano e che chi governa abbia il dovere di pesare le parole più di chiunque altro. La minaccia di chiudere i porti italiani aveva chiaramente lo scopo di esercitare una pressione, ma che purtroppo si è rivelata inutile sugli altri Paesi europei. Ma in Italia anche questa ha contribuito ad alimentare paure e fobie che, al contrario, chi governa ha il dovere di contenere e stemperare. L'offensiva contro le ONG che si sta preparando avrà lo stesso effetto, moltiplicato. Siamo certamente di fronte a una situazione difficile, determinata più dall'egoismo dell'Europa che dal flusso migratorio. Ma non siamo di fronte a nessuna invasione enorme. Non possiamo continuare ad alimentare l'idea dell'invasione. In Africa, certo, è in corso un gigantesco esodo di popolazioni che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalla carestia, ma i dati chiariscono le reali dimensioni del fenomeno: solo un quinto un quinto di questo esodo di massa si dirige verso l'Europa, e solo il 2,5 per cento di chi muove verso l'Europa lo fa passando per l'Italia. Non significa che si debbano chiudere gli occhi, ma certo dobbiamo assolutamente evitare di rincorrere le forze xenofobe sul loro terreno e di fomentare l'allarme sociale, perché questo non aiuterà questo non aiuterà a risolvere niente; renderà solo tutto molto più barbaro e anche noi un po' più barbari.

come se lei e il suo Governo vi foste insediati oggi. Ma, Ministro, il suo tentativo non funziona perché i responsabili di questa emergenza hanno un nome e un cognome.

Per mesi lei ha fatto credere al Paese che il Governo stesse facendo fronte a questa emergenza, ma i numeri la smentiscono clamorosamente:

cioè immigrati da rimpatriare e non profughi di guerra o perseguitati che fuggono da dittature. Questi dati certificano il fallimento del Governo Renzi, del PD che l'ha sostenuto e del suo Governo, ministro Minniti, soprattutto, il fallimento di un'idea di un'Europa solidale, che si è miseramente infranta sulle barriere che hanno alzato Paesi come la Francia, la Spagna, l'Austria, i nostri vicini. Per mesi avete accusato il Movimento 5 Stelle di populismo, addirittura in taluni casi di razzismo, solo perché abbiamo osato proporre soluzioni di buonsenso, buonsenso, che avete tentato di ascrivere a un'ideologia, a volte di sinistra, a volte di destra, per poi dover riconoscere che le nostre proposte erano evidentemente sensate, al punto tale che oggi le avete fatte vostre e andate addirittura a presentarle in Europa. Vediamo queste proposte. Il Movimento 5 Stelle, sin dal 2014, ha chiesto di rivedere gli accordi di Dublino III e di ridistribuire le quote di migranti negli altri Paesi, sanzionando gli Stati membri che non collaborano. Oggi lo chiedete anche voi. Ma io mi chiedo: chi ha siglato, Ministro, gli accordi di Dublino luogo, abbiamo chiesto di rivedere Triton, l'operazione che autorizza le navi di 15 Stati europei a raccogliere e portare i migranti solo in Italia.

Inoltre, nei giorni scorsi l'ex ministro Emma Bonino ha dichiarato che è stata l'Italia, con il PD al Governo, a decidere di accogliere tutti gli immigrati. Le chiediamo: in base a quali accordi, visto che una cosa del genere non è mai stata ratificata dal Parlamento italiano? Il Movimento 5 Stelle per primo ha lanciato l'allarme sulle operazioni di salvataggio dei migranti ad opera di alcune organizzazioni non governative internazionali. Lo abbiamo fatto dando voce all'allarme lanciato da un procuratore della Repubblica. Abbiamo proposto di chiudere i nostri porti a quelle ONG che non hanno bilanci trasparenti e che spesso battono bandiera di Paesi paradisi fiscali. Ci avete accusato di incompetenza e poi, a distanza di qualche mese, voi stessi avete minacciato l'Europa dicendo che avreste chiuso i porti alle ONG e alle imbarcazioni che non rispettano le regole, invocando una regolamentazione per queste organizzazioni. Simeoni)*. Abbiamo presentato un disegno di legge per consentire alle procure di poter compiere le indagini anche in mare aperto e, soprattutto, sulle navi delle ONG. E oggi lei cosa viene a dirci?

Siamo costretti a gioire per alcune elemosine dell'Europa, perché di questo si tratta: i 35 milioni di euro sono un obolo con cui l'Europa si lava la coscienza;

dei 10 miliardi che l'Europa - e quindi anche l'Italia - ha dato alla Turchia per proteggere la Germania dal flusso migratorio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tra l'altro, quei 10 miliardi hanno ulteriormente aggravato il carico sulla rotta mediterranea e quindi gli afflussi nel nostro Paese. Questi soldi, così come le frontiere chiuse di Francia e Spagna e la minaccia dell'esercito al confine del Brennero, sono uno schiaffo in faccia al nostro Paese, una presa in giro che un Governo serio e autorevole non dovrebbe accettare. Gentiloni Silveri, invece, "apprezza". Ma come fa ad apprezzare? Questi 35 milioni sono veramente briciole. I traffici degli esseri umani fanno gola a chi vuole alimentare il *business* dell'accoglienza e a tutti coloro che, grazie alla complicità di una buona parte della politica, lucrano sulle emergenze migratorie. Questa situazione è insostenibile e intollerabile e la responsabilità è sua e di questo Governo. Occorre cambiare passo, signor Ministro, in Italia e soprattutto in Europa. Altrimenti, il rischio sarà quello di far precipitare il nostro Paese in quella che sembra sempre più essere

Signora Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il ministro Minniti per avere riconosciuto a questa Camera e, in particolare, alla Commissione difesa, il lavoro svolto con questa indagine conoscitiva che, lo voglio ricordare, è stata provocata anche da una nostra richiesta.

sono alla base del documento con il quale abbiamo lavorato a Parigi e che, probabilmente, potrebbero essere anche la base per un lavoro comune con l'Europa. Io vorrei partire dalla fine del suo intervento, signor Ministro. Lei ha detto:

che l'accoglienza aveva, e secondo lei ha, un limite nella sensibilità del Paese. Lei ricorderà queste parole. Io apprezzai questo passaggio, perché non vi è solo un problema di limite alla capacità di integrazione, ma vi è un limite che risiede nella sensibilità del nostro Paese. Infatti, lei ha proseguito oggi nel suo intervento dicendo che è in gioco la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese. Questa è una frase importante, perché vuol dire che sta succedendo qualcosa nel nostro Paese, per cui c'è il rischio che il tessuto connettivo delle nostre città, delle nostre famiglie e delle nostre piazze non tenga più.

Il ministro Minniti ha detto a tutti noi: attenzione, è cambiato il mondo dell'immigrazione non regolata. Fino a due anni fa, sulla rotta balcanica vi era una immigrazione di rifugiati e richiedenti asilo che venivano dalle zone di guerra; oggi, siamo di fronte a migranti economici. Il *push factor* che sta nascendo, che è nato nei Paesi della fascia subsahariana si è totalmente e completamente sostituito dei rifugiati, delle famiglie e di coloro che scappano dalle guerre della Siria, dell'Iraq e dell'Afghanistan. Quel fenomeno non esiste più. La rotta balcanica si è prosciugata e non solamente perché la Turchia tiene tre milioni di rifugiati siriani. Peraltro, di quei tre milioni, signor Ministro, forse lei sa che 500.000 sono già tornati in Siria. Sono tre milioni di persone che non hanno voglia di venire in Europa, se non per scappare dalla guerra, ma hanno solo voglia di tornare nei loro Paesi: perché quello è il loro Paese, quella è la loro storia, quelle sono le loro tradizioni. L'Europa ha stanziato 3 miliardi e ha consentito alla Turchia di tenerli e di farli sopravvivere in campi che sono sicuramente più decorosi di quelli che ci sono in Libia. Ma quello è stato un fenomeno,

lei oggi, in esordio di intervento, ha parlato di ventiquattro navi al limite delle acque territoriali a raccogliere coloro che andavano sì salvati, ma per il fatto stesso che erano lì, quello era comunque un fattore di attrazione per coloro che fuggono dalle spiagge libiche. oggi nel suo intervento, proprio nella distinzione che ha voluto fare, ha anche detto che che c'è un problema di ricollocazione, che però è inesatta come definizione per quanto riguarda i migranti economici. Nel 2015, il Consiglio europeo ha parlato sì di ricollocazione, ma lo ha fatto con un documento nel quale alla fine si era detto che la ricollocazione poteva avvenire, secondo certe quantità, sulla base di una soglia definita del 75 per cento, che era la media statistica dell'accoglimento delle richieste di asilo rispetto ai Paesi da cui si fuggiva; e se non si superava quella soglia, le ricollocazioni non erano consentite. Ma si parlava con esattezza solo di rifugiati, solo di richiedenti asilo. Il fenomeno con il quale oggi abbiamo a che fare è totalmente diverso: parliamo di migranti economici. E Macron cosa ci ha detto? Se si parla di richiedenti asilo, siamo disponibili anche ad ampliare le quote, ma voi avete i migranti economici; voi avete un altro fenomeno e noi non siamo disponibili ad accoglierli. Quindi, ribadisco, è cambiato il mondo e con questo drammatico cambiamento abbiamo a che fare. Qual è allora la terapia?

ma forse era più giusto farlo qui: lei ha detto anche che potrebbero essere riportate in Libia le persone che vengono salvate. Ciò vuol dire che anche il nostro Governo comincia a pensare che ci possa essere la possibilità di intercettare coloro che salpano - mi perdoni: potremmo anche evitare che salpassero, ma ammettiamo pure che possano salpare - e, in collaborazione con le autorità locali (non meglio definite, perché tutti sappiamo che non abbiamo un'unica guardia costiera libica, bensì tre), potremmo riaccompagnare, come in diecimila casi è avvenuto, coloro che sono partiti, senza che affondino, senza che anneghino, senza che muoiano a poche centinaia di metri dalle coste libiche. Ciò vuol dire che per questo Governo - e questa è anche una domanda, ma avremo tempo per parlarne e discuterne - l'unico piano B - non c'è più il presidente Casini, ma a questo immagino alludesse alludesse - possibile e immaginabile per risolvere il problema dei migranti economici è che non partano. Non si può più partire dalle coste libiche. Se è vero quello che dice

nei prossimi anni, secondo voi è mai ammissibile che nel nostro Paese possano arrivare, in un modo o nell'altro, 295.000 persone che vengono in Italia e in Europa solo per un problema di carattere economico, solo perché il Sud del mondo sta premendo sul Nord del mondo?

ad utilizzare lo strumento militare, che pur costa 30 miliardi all'anno e che forse varrebbe anche la pena di utilizzare laddove ce ne fosse la necessità - di utilizzare lo strumento militare,

all'UNHCR. Vuol dire che non vengono controllati dalle organizzazioni internazionali, bensì sono nella possibilità di ricevere le visite di organizzazioni internazionali. Allora, vuol dire che ci sono dei campi che si potrebbero rafforzare, alcuni addirittura sono sotto il controllo del Governo Serraj che, a quanto mi constava, era rifugiato nel porticciolo di Tripoli. Forse, invece, riesce ad avere anche un minimo di apertura. Forse quel MOU (Memorandum of undestanding) che lei, Ministro, ha fatto con il Governo Serraj può comprendere anche il controllo, l'accesso,

di venire in Italia possono essere messe nelle condizioni di rimanere là dove si trovano adesso, in condizioni migliori grazie alle organizzazioni internazionali, grazie anche alla nostra collaborazione. davvero dicendo forse una cosa che non tutti sanno. A Mosul, come sapete, stanno conquistando la cittadella antica: sono poche centinaia di metri quadri ormai. Sapete che intorno alle mura di quella cittadella ci sono i corpi speciali francesi e inglesi? Secondo voi che cosa fanno? Intercettano i *foreign fighter*. Il termine «intercettare» comprende qualsiasi tipo di significato in una guerra moderna: significa che questi due grandi Paesi - come è grande il nostro - si mettono nelle condizioni di evitare che questi criminali tornino nei Paesi d'origine. Bene, Ministro, forse qualche pensiero al riguardo, per evitare che qualche criminale di troppo giri, si agiti e faccia i suoi sporchi affari sul territorio libico, Signor Ministro, innanzitutto mi permetta di ringraziarla non soltanto per il lavoro che sta facendo in questi mesi, ma anche per aver ritenuto necessario venire a svolgere questa sua informativa alle camere, a testimonianza della considerazione che ha del Parlamento; valore, questo, che, in questo periodo, di questi tempi, ha un significato particolare. Come lei ha sottolineato, siamo di fronte a un fenomeno di portata epocale. Io sono francamente colpito, molto spesso, dal semplicismo con il quale si sta trattando una materia che ha una portata enorme. Mi hanno insegnato che uno degli ingredienti fondamentali per decifrare anche i fenomeni profondi

della popolazione nei prossimi anni, fino al 2050, sarà di circa 4 miliardi, metà dei quali saranno tutti concentrati in Africa. Dunque, questo fenomeno, con il quale noi - mondo - dobbiamo abituarci a fare i conti nei prossimi anni, deve essere affrontato senza sciocche semplificazioni e ben sapendo che la soluzione della crisi migratoria non è dietro l'angolo. Occorre avere questa consapevolezza e l'approccio che lei ci ha proposto, con la svolta che è stata introdotta con questo approccio, e cioè di passare dal misurarsi con questo tema in una chiave emergenziale al misurarsi in una chiave strategica, è il passaggio fondamentale per poterci misurare nella maniera migliore possibile con questo Gli ingredienti di questa prospettiva strategica - lei li ha descritti nella sua comunicazione - sono molteplici e tutti devono essere in sintonia tra di loro, a partire da un'iniziativa che assume il tema della stabilizzazione della Libia come *asset* centrale. centrale. In questo senso, caro collega Romani, lei sa quanta stima io abbia delle sue considerazioni, ma noi abbiamo fatto una scelta: quella di rendere il popolo libico protagonista di questo processo, dunque di evitare di ricommettere quegli errori che abbiamo commesso nel passato e che hanno prodotto la situazione con la quale stiamo facendo i conti, prevedendo, certo, anche l'impegno di energie militari militari a supporto di un'azione di stabilizzazione, di un'azione di *training* e di formazione, come sostanzialmente si sta facendo.

quello di un lavoro che non rinuncia all'assoluta esigenza di salvare le vite umane, un principio irrinunciabile, quello di procedere a politiche di gestione dei flussi migratori che accolgano coloro i quali hanno diritto ad essere accolti e, garantendo il rispetto dei diritti delle persone, producano il rimpatrio di quelli che non hanno diritto all'accoglienza. Sono tutti ingredienti ed in questa cornice si colloca anche il ruolo delle organizzazioni non governative: o il loro è un ruolo inserisce in un'attività strategica di questa natura e dunque è funzionale a gestire complessivamente il fenomeno, altrimenti sono stupito dalle dichiarazioni di alcuni esponenti delle ONG, perché in nessuna parte del mondo in cui le ONG operano ed hanno un ruolo fondamentale possono agire in conflitto, in questo caso con il Paese che indica la prospettiva strategica entro cui si colloca. In questo quadro, il tema è rendere gestibile l'insieme delle questioni e, in questa fase, mi permetto di dire di rendere gestibile una peculiarità con la quale stiamo facendo i conti in questi giorni, che non è soltanto la dimensione quantitativa del fenomeno, ma è anche l'aspetto della sua temporalità: soltanto in un *weekend* sono soltanto in un *weekend* sono arrivate 12.000 persone e ne arrivano ogni giorno e questo mette a dura prova non soltanto la capacità di risistemazione, di ridefinizione e di governo di queste quantità, ma persino il lavoro delle nostre Forze dell'ordine, che, come sapete, in ogni situazione di questo devono certificare l'aspetto sanitario, devono identificare i singoli e devono avviare quelle procedure che poi, via via, devono essere seguite per poter gestire la situazione nei termini che sono stati sopra descritti. Questo è il tema che abbiamo di fronte e in questo quadro è chiaro che tutto si deve coniugare ad una irrinunciabile battaglia

dunque si deve tenere ed il tema cruciale è quello di tenere insieme tutto questo con le politiche di integrazione, facendo tesoro, peraltro, del fallimento delle politiche di integrazione che altri Paesi hanno condotto (penso alla Francia o alla Gran Bretagna), quindi dobbiamo anche definire un nuovo modello di integrazione, diventare quasi un Paese laboratorio da questo punto di vista. Tutto si deve tenere e laddove uno di questi ingredienti viene meno, salta quell'equilibrio che è l'unico modo per misurarsi con questo problema e per garantire la tenuta della democrazia, i principi di sicurezza, la tutela della dignità umana. Se uno di questi ingredienti non funziona, inevitabilmente andiamo in difficoltà. Il lavoro che stiamo facendo e che lei sta facendo, signor Ministro, e che noi ci sentiamo di poter dire che intendiamo supportare, continuando questo rapporto tra Parlamento ed Esecutivo, che diventa ingrediente anch'esso fondamentale di questo lavoro, va in questa direzione. L'Europa, come ha detto il Presidente del Consiglio, in questi anni ci ha voltato le spalle. Questa iniziativa non sta determinando ancora un cambiamento radicale dell'atteggiamento europeo, però, mentre fino a ieri le porte ci venivano sbattute in faccia, ora si cominciano ad aprire. Facciamo non trascurare i pur piccolissimi ed insufficienti passi in avanti che da questo punto di vista si stanno facendo, perché è su di quelli che poi dobbiamo costruire la nuova fase della nostra iniziativa e quello di domani, a Tallin, è un incontro informale (vale la pena ricordarlo), cioè sarà un'occasione per approfondire questa discussione e per predisporsi anche a creare ulteriori condizioni perché dalle parole si passi ai fatti. Sarà importante,

per portare avanti questa iniziativa e raggiungere degli obiettivi. Se invece qui dovesse prevalere la tendenza a esasperare la polemica politica, con il miope obiettivo di incassare qualche consenso in più,